Comunico che in data 21 settembre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali,

L'artista si ricollega indissolubilmente all'uomo; più è importante la ricchezza dell'uomo, più sarà profonda quella dell'artista dirà il compositore Marij Kogoj. Aldo Daneu Danieli è stato un cosmopolita, ma anche un uomo fortemente legato alla sua terra, al Carso. Un grande talento, il suo, che lo ha condotto da Trieste, dove si è formato musicalmente musicalmente al conservatorio Tartini, a dirigere nei più importanti teatri lirici del mondo, da San Francisco alla Fenice di Venezia, al coro dell'Arena di Verona e al teatro Colón di Buenos Aires, lavorando come maestro collaboratore con l'opera di Vienna, della sua Trieste, di Napoli, Palermo, Torino, con numerosi teatri in Germania e con grandi artisti della lirica che con lui approfondivano e perfezionavano la tecnica vocale e si preparavano ad affrontare importanti ruoli operistici. Tra tutti, vorrei ricordare la grande amicizia e la *liaison* artistica col tenore Carlo Cossutta, indimenticabile interprete interprete verdiano di fama mondiale. Il maestro Danieli si vide italianizzare il proprio nome - nasce infatti sloveno, come Adi Daneu - e al suo definitivo rientro a Trieste volle dedicarsi alla propria comunità. Compositore e interprete raffinato di molte pagine operistiche, anche di autori contemporanei, aveva pubblicato un libro dedicato alla tecnica vocale, che veniva spiegata con minuzia e sapere, ma intrisa di aneddoti della sua lunga vita artistica come pure da caricature e disegni coi quali amava raccontarsi. Ha voluto sfidare se stesso nella convinzione che non esistono limiti alla capacità di un gruppo di cantori di interpretare la musica, preparando corali di amatori ed esibizioni di grande intensità. Una guida sapiente, un artista a tutto tondo con uno spessore culturale tale da permettergli anche sfide artistiche impensabili. Amabile conversatore, seguiva la politica e la cultura e ne amava disquisire pur sedendosi al pianoforte. Uomo di grande ironia e semplicità, insignito di importanti riconoscimenti tra i quali quello di Cavaliere della Repubblica. Ho avuto l'onore di collaborare con lui più volte e di scrivere la nota introduttiva del suo già citato volume. Rimarrà di lui il sapere che condivideva con grande generosità, la sua autoironia, la sua galanteria, ma soprattutto il lavoro che rende indelebile il suo ricordo. Ai suoi familiari, ai suoi allievi e agli amici un commosso abbraccio. Ciao maestro,

le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano sono una componente fondamentale dell'affermazione del *made in Italy* sui mercati globali, e il sistema europeo delle indicazioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela. Grazie alla distintività della nostra produzione, l'Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti: sono 838 le DOP e le IGP iscritte. L'Italia non produce cibo: l'Italia produce distintività, cultura e tradizione. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre 180.000 addetti, per un valore della produzione pari a circa il 20 per cento del totale agroalimentare nazionale. Oggi la ripresa del settore agricolo e della trasformazione industriale dipende in larga parte dalla crescita del mercato estero, e i primi dati di quest'anno indicano che nel 2021 potrebbe essere superata la soglia storica di 50 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari: un risultato davvero eccezionale per i nostri produttori. È pertanto necessario potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che costituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi. Una tutela che passa anche attraverso la lotta alla contraffazione del cosiddetto *italian sounding*, ambito in cui l'attenzione del Ministero è sempre elevata grazie alla costante ed efficace azione di controllo dell'ispettorato e del comando Carabinieri per la tutela agroalimentare. All'interno dei marchi a denominazione, il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi anni. Nel 2020 sono state prodotte 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo: un dato che parla da solo. Nell'arco di poco più di un decennio dalla sua costituzione, il 2009, il Prosecco è diventato la prima DOP italiana del comparto del vino. Negli ultimi cinque anni, sia le esportazioni che il valore della produzione sono aumentati di circa il 30 per cento, arrivando a sfiorare una quota del 25 per cento del valore totale nazionale delle DOP del vino. Nello stesso periodo di tempo il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella crescita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una quota di oltre il 16 per cento del totale. È del tutto evidente che il prosecco traina tutto il settore agroalimentare. Oggi i tre quarti delle bottiglie prodotte sono collocati all'estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati dell'*export* di vino del primo semestre 2021, come dicevo prima, che cresce del 15,2 per cento rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2 per cento del settore agroalimentare nel suo complesso. È anche per tali ragioni che alla vicenda oggetto dell'informativa odierna, che vado a ricostruire, è rivolta la massima attenzione da parte mia e del Ministero, al fine di tutelare il mercato agroalimentare italiano e una delle nostre eccellenze vitivinicole. Nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all'attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek del settore vitivinicolo presentata dalla Croazia, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento UE n. 1308 del 2013. Sin da subito, già nel corso del Comitato di gestione europeo del 29 giugno, abbiamo espresso la netta contrarietà alla proposta in quanto, non solo la traduzione di detta menzione corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli asolani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione, ma anche perché - e voglio sottolinearlo con forza - l'eventuale autorizzazione all'uso del Prošek croato avrebbe creato e creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'*italian sounding*. Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda e, pur mantenendo ovviamente altissima l'attenzione sulla vicenda, tengo a rassicurarvi sul fatto che ad oggi non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prošek, dal momento che la normativa europea ci consente, in sede di opposizione, di fare valere le nostre ragioni. Ad oggi la Commissione ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della domanda. Tutta la fase di merito sarà lunga e seguirà a questo percorso.

nell'asserire che la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell'Italia sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt'altro che conclusa e, in una riunione con gli assessori a margine degli eventi del G20, ha dichiarato espressamente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire. Come previsto dalla normativa europea, dunque, nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di registrazione in *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione ad oggi non ancora intervenuta) faremo opposizione formale nei confronti della domanda croata e lo faremo in modo adeguato e compatto, sia con l'ausilio delle strutture tecniche del Ministero, sia con la pressione, l'azione e l'interlocuzione politica che eserciteremo nei confronti di Bruxelles. È già stato attivato, infatti, un tavolo tecnico per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità, al fine di opporci a quanto proposto dalla Croazia.

e che, anzi, in virtù della sua delega oggi ha voluto essere presente proprio per rappresentare l'unità del Governo e di come ci muoviamo in modo sincrono - sin da subito ha attivato appunto un *dossier*, anche in ragione della sua delega. lui ho personalmente chiesto di agire assicurando il coordinamento necessario a rendere proficua ed efficace l'azione ministeriale nel suo complesso. Ci sono molti argomenti a sostegno delle nostre ragioni, che mi fanno ben sperare sul lieto fine della vicenda, che festeggeremo stappando un'ottima bottiglia di Prosecco, posto che in ogni caso, non essendo ancora intervenuta la pubblicazione della domanda da parte croata, gli elementi informativi di cui disponiamo sono necessariamente limitati. Non conosciamo ancora il merito e il contenuto della domanda, ma ovviamente la analizzeremo nel dettaglio appena pubblicata in Gazzetta. Rilevo, infatti, che un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prošek si pone in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 e non è questo il caso. A tal riguardo, ricordo che già dai negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte della Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta in tal senso e, su opposizione dell'Italia, tale richiesta venne respinta. Infatti, la menzione tradizionale Prošek non venne iscritta nel registro della Commissione UE. Ci appelleremo inoltre a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso 9 settembre nell'ambito della causa C-783/19 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB, nota anche come sentenza Champanillo), vale a dire che sussiste evocazione abusiva quando «l'uso di una denominazione produce nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall'intercorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra DOP e la denominazione di cui trattasi o, ancora, da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione». Ebbene, non spetta a me dirlo, ma appare indubbiamente come il termine Prošek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il prosecco italiano. Peraltro, non esiste un paese che si chiami Prošek, mentre esiste una località nel Comune di Trieste che si chiama Prosecco. Pertanto, ritengo che non ci siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato. Se ciò avvenisse, infatti, verrebbe palesemente smentito un autorevole principio giuridico affermato dalla Corte di giustizia europea e recentemente ribadito. Ho già sottolineato quanto sia grande, forte e importante la produzione di Prosecco per il nostro sistema agroalimentare e vitivinicolo. A questo settore ribadisco l'impegno mio e di tutto il Governo a mettere in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata ed assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i produttori e consumatori. Auspico vivamente - ma ne sono più che convinto, vista anche la richiesta di informativa di avere il supporto di tutti voi, oltreché dell'intero Governo, per quella che necessariamente non può che essere una battaglia di tutto il nostro sistema Paese a favore di una delle sue più importanti e distintive eccellenze.

per il suo dichiarato impegno e il Sottosegretario per il lavoro che già è stato fatto in queste settimane su questo tema. Credo che oggi in questa un sostegno forte e unanime da parte di tutto il Parlamento, che interpreta - penso in modo adeguato - il sentimento del Paese. Ritengo non vi siano dubbi sul fatto che questa battaglia (così la chiamo) sia fondamentale

produzione vitivinicola, più di 10.000 aziende agricole e 1.500 tra case vinicole e spumantiere, che interpretano un sistema economico straordinario che è la prospettiva e il futuro del territorio, ma anche uno degli ambasciatori e vessilli della qualità del *made in Italy* nel mondo. Da questo punto di vista credo che tutti insieme porteremo avanti questo tipo di impegno e questo tipo di battaglia. Mi permetto però di sottolineare che qui non è in gioco soltanto il futuro del prosecco e del suo territorio, ma è in gioco un modello di tutela alimentare, che è quello delle denominazioni di origine che l'Unione europea si è data e di cui, come diceva giustamente il Ministro, l'Italia è il Paese protagonista assoluto con oltre 800 specialità garantite e certificate che dichiarano al mondo il proprio modello produttivo, la propria storia, le proprie tradizioni, che definiscono gli ambiti territoriali nei quali queste produzioni vengono realizzate. È in gioco un modello che è un patrimonio culturale, che è la salvaguardia di territori e di comunità. Credo che sia evidente a tutti che in questa stagione questo modello è sotto attacco, come la vicenda dell'aceto balsamico delle scorse settimane testimonia. Ritengo inoltre che a testimoniarlo vi siano una una molteplicità di iniziative che tendono a mettere in discussione questo modello, che dal nostro punto di vista è fondamentale perché garantisce trasparenza ed autenticità nei confronti dei consumatori, tutela di tradizioni culturali che sono fondamentali per determinati territori. A tale riguardo la battaglia e il nostro impegno a difesa di tale modello culturale e la richiesta all'Unione europea

difesa del nostro modello Prosecco, è la difesa del consumatore, come rilevato bene dal Ministro. C'è l'evocazione di un nome, peraltro su un vitigno e su un vino che è fermo e non c'entra nulla con l'idea del Prosecco, che se approvato, rischierebbe di ingenerare nel consumatore un'assoluta confusione su quello che è il prodotto di cui trattasi. Da questo punto di vista la riflessione che ci portava il Ministro sul concetto di evocazione credo sia straordinariamente importante proprio perché è un «baluardo» di difesa del diritto del consumatore per sapere cosa sta comprando. Ecco, visto che i minuti passano veloci, mi permetto di riassumere sostanzialmente

Noi abbiamo tutti gli elementi per dire e per muoverci a difesa di un prodotto avendo, dal nostro punto di vista, tutti gli elementi giuridici per poterlo fare. una battaglia anche politica; noi dobbiamo stringere sempre di più alleanza con tutti quelli che credono nel nostro modello produttivo incentrato sulle denominazioni di origine, perché questa è una battaglia che giochiamo oggi, ma che giocheremo in futuro se vogliamo tutelare il nostro modello alimentare. È altresì una battaglia culturale sul modello di agricoltura, sulla difesa dell'autenticità e la non massificazione dei prodotti.

battaglia rimane solo italiana, rischiamo di perderla; se diventa una battaglia che vede nell'Italia l'alfiere dell'Europa e di tutti coloro che nel mondo credono in questo modello, possiamo vincerla e per i consumatori questa sarà una scommessa fondamentale.

delle eccellenze italiane. Lei, signor Ministro, ha ricordato opportunamente i numeri: quest'anno si raggiungeranno nell'agroalimentare i 50 miliardi di esportazioni, che sono una fetta significativa e importante. Io sono un convinto europeista, da sempre,

l'idea che si possa prendere un vino che assomiglia al nostro è contro il livello istitutivo delle nostre denominazioni europee.

secondo luogo, io vengo dall'Est veronese dove c'è una denominazione che si chiama Soave e identifica un paese, quello di Soave. Pertanto non può esserci nel mondo qualcun altro che brevetta o deposita un marchio con quel nome, perché veramente faremmo dei disastri assolutamente incalcolabili. Questa richiesta della Croazia dell'iscrizione nelle DOC del Prosecco sta già creando, secondo i dati ufficiali del consorzio del Prosecco, gravi danni danni in termini di esportazione: già oggi questa situazione sta creando un danno nella nostra prima eccellenza di esportazione nell'ambito dell'agroalimentare. L'autorizzazione al Prošek creerebbe un precedente pericoloso: considerate che i nostri principali alleati in questa battaglia saranno i francesi dello Champagne e gli spagnoli, perché si introduce un *vulnus* veramente pericoloso. È in pericolo la credibilità europea anche nei confronti dei Paesi terzi, specialmente nel mercato americano dove, anche se il Prosecco è il primo in termini di fatturato, la penetrazione commerciale non è ancora forte. Si tratta, quindi, di una battaglia

Signor Ministro, lei ha detto che il Governo c'è tutto, dica al presidente Draghi che su questa questione non si può arretrare di un centimetro; dobbiamo tenere una posizione

Già oggi ci sono risultati negativi nelle vendite, specialmente nel mercato nordamericano. Io non so come saranno le procedure, ma a qualsiasi livello di negoziazione su questa questione, signor Ministro, signor Sottosegretario, signori del Governo, va posta una difesa della nostra bandiera. avanti, non molliamo e sicuramente avrete l'appoggio incondizionato di tutto il Parlamento e anche di Forza Italia.

con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per il riconoscimento del Prošek*.* Sebbene la parola Prošek sia molto simile allo spumante italiano prosecco poi non ci sono sono somiglianze tra i prodotti, né per il metodo di produzione, né per lo stile, né per le uve utilizzate. Non c'è alcuna relazione neanche tra le origini dei due nomi. Il Prošek, lo sappiamo, è un vino tradizionalmente dolce, da *dessert*, proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia. Si tratta, quindi, di un prodotto completamente differente dal Prosecco italiano che, invece, è fiore all'occhiello della produzione vitivinicola italiana, che abbraccia due Regioni, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, Province e tre denominazioni d'origine: Prosecco Doc, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Asolo Prosecco Doc, per una produzione complessiva che ha superato 600 milioni di bottiglie, dopo aver incassato, nel 2019, l'importante riconoscimento dell'Unesco per le colline del Prosecco. La Cia di Treviso ha sottolineato in queste settimane come i grandi risultati conseguiti dalle denominazioni di Prosecco, proprio grazie al duro lavoro e alla determinazione di generazioni di viticoltori, siano oggi in grave pericolo. Si sta assistendo a una gravissima violazione dell'identità di una comunità e di un territorio che si riconosce in una produzione enologica di grande eccellenza. Per questo, come senatrice di Italia Viva, soprattutto per il legame che ho con il mio territorio, con il Veneto, sento particolarmente vicino l'appello delle associazioni di categoria affinché ci si adoperi, in ogni sede e tavolo, per tutelare le nostre produzioni agroalimentari. Desidero qui, in Senato, esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto da tutte le associazioni di categoria, a livello provinciale, regionale e nazionale, perché è a fianco dei consorzi e dei produttori dobbiamo stare tutti uniti, a difendere le nostre produzioni agroalimentari e tutelare un intero comparto che tanto valore sta portando all'Italia e ai nostri territori. Ci troviamo ancora in una fase prodromica della vicenda, ma per questo occorre, in tempi rapidi, fare fronte compatto, tutti quanti, per un'opposizione adeguata ed efficace. In questo senso, mi fa ben sperare ciò che lei, signor ha già detto, nelle scorse settimane, ma soprattutto nel suo intervento di oggi: il lavoro fatto dalle associazioni di categoria deve trovare una sponda robusta nelle istituzioni e nel Governo per poter ottenere dei risultati apprezzabili. Dobbiamo fare quadrato per salvaguardare un'eccellenza del nostro Paese. Io non voglio citare, perché l'ha fatto già lei, le recenti decisioni della Corte di giustizia europea, europea, ma la decisione della Commissione europea, questa sì, ci lascia alquanto perplessi. Noi dobbiamo difendere i nostri prodotti. Non sarà un percorso facile né semplice, perché il Prošek non è una banale imitazione delle più ben note bollicine venete e friulane. Ha una storia alle sue spalle, certamente, ma la convivenza tra i due prodotti è sostanzialmente impensabile. Ha ricordato bene anche lei cosa tale convivenza genera sui mercati internazionali. Parliamo di una bollicina italiana che oggi supera le 620 milioni di bottiglie, con un fatturato complessivo di 2,4 miliardi, di cui il 78 per cento all'estero. Anche per questo la decisione della Commissione europea è un precedente pericoloso, che rischia di indebolire la stessa Unione europea

sull'aspetto della confusione che si potrebbe generare, dato che è proprio il consumatore che fa la differenza nel successo di un prodotto. Qui non possiamo permetterci errori. Non è sufficiente leggere le etichette o notare le differenze di luogo o di produzione, perché è molto semplice che una parola assonante diventi molto rapidamente identitaria nell'immaginario collettivo. Noi su questo dobbiamo essere molto fermi tutelare i consumatori, tutelare ed essere a fianco e sostenere gli operatori agricoli, il territorio e la qualità della denominazione Prosecco. Una storia, una tradizione, una cultura, la cui notorietà, ormai consolidata in tutto il mondo, non può essere sfruttata a vantaggio di altri. Dobbiamo quindi agire rapidamente, signor Ministro, - come ha appena detto - perché abbiamo a disposizione pochi giorni, proprio dalla data di pubblicazione, per presentare un'obiezione che la Commissione europea analizzerà prima di adottare una decisione finale. Fortunatamente - ne sono dimostrazione oggi gli interventi che mi hanno preceduta si tratta di un tema trasversale: Governo, associazioni di categoria e noi rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli siamo tutti chiamati a fare fronte comune per predisporre un'azione rapida, efficace e adeguata. Diventa quindi ancora più fondamentale che ci si muova in maniera compatta. Va condiviso un comune percorso di intenti che ci permetta di presentare obiezioni forti alla Commissione europea, così da scongiurare non solo un attacco al nostro Prosecco, ma a tutto il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo.

e di una denominazione storica, come quella rappresentata dal Prosecco. D'altra parte, qualsiasi differente scenario finirebbe per svuotare di ogni significato la nozione stessa di DOP e, in definitiva, sconfessare i valori fondamentali che gli Stati membri e la stessa Unione europea sono chiamati a perseguire. Ciò finirebbe per creare un precedente che parzialmente minaccerebbe tutte le denominazioni europee e le eccellenze tutelate.

opporsi con ogni mezzo a questo riconoscimento che rischia di arrecare un notevole danno economico a uno dei prodotti di punta del *made in Italy* agroalimentare. Signor Presidente, ringrazio il Ministro ed esordisco subito con una brutta notizia. È di questa mattina la presentazione da parte

abbastanza ben visto da questa parte politica - mi sembra evidente - perché la maggior parte delle volte in cui è venuto in quest'Aula ha chiesto di difendere i prodotti nazionali, qualche volta trascinato da noi, come sulla questione nutri-score, prima alla Camera e poi al Senato, e anche oggi, con questa informativa sul Prosecco, che condivido debba essere un tema di assoluta trasversalità

Sinceramente, non è che questa Nazione - non per colpa sua, ma anche di chi l'ha preceduta - oggi abbia un piano per l'agricoltura nazionale che possa dirsi fattore di sviluppo e di aumento dell'*export.* Lavoriamo su questo, noi siamo a disposizione. Come abbiamo sempre detto, quando c'è da costruire, ci troverete sempre al vostro fianco. Rigettiamo anche le critiche nei confronti dei Ministri che non sono competenti per materia,

all'interno di un terreno agricolo, quindi avremmo dovuto arrabbiarci tutti nei confronti di quell'orgia di illegalità che è avvenuta in Provincia di Viterbo. Non vorrei che, per lo stesso principio per cui in Italia è concesso tutto,

abbiamo raggiunto i 100 miliardi di prodotti copiati, quindi è evidente che sono in atto, come per il nutri-score, una forma di discriminazione nei confronti dei nostri prodotti e un tentativo di erodere i nostri mercati.

- le chiediamo di fare un gruppo di lavoro all'interno del suo Ministero che si occupi di questo tipo di difesa, facendosi aiutare anche dall'avvocatura.

un'unità di intenti e una compattezza che non ci facciano percepire come la cenerentola d'Europa: oggi accade per il Prosecco, domani accadrà per il nutri-score*,* dopodomani per qualsiasi altro prodotto che si intenda svilire. Se non lo facciamo, siamo costantemente in difesa.

che non riescono mai a fare programmazione, semplicemente per il fatto che devono perdere tutto il loro tempo a difendersi dalle accuse, dalle responsabilità, a volte da un Governo ostile - dai tanti che lo sono, non solo questo questo - che vede i piccoli Comuni quasi come il male assoluto. Ecco, vorremmo che fosse liberato da queste incombenze e potesse

che oggi vede i maggiori aumenti nell'*export*, non sono del vino: da 670 milioni di bottiglie a 370 milioni di *export*; il Prosecco da solo vale 2 miliardi,

signor Ministro, mi sembra che dalla discussione di questa mattina stia emergendo in maniera plastica l'importanza della produzione del Prosecco nel nostro Paese. I tre consorzi capofila hanno creato un prodotto di qualità: certo, potremmo anche discutere della qualità differenziata a seconda di dove viene prodotto e della tipologia di produzione, ma certamente di qualità;

Quando parliamo di questo, sappiamo di cosa stiamo parlando: l'Italia, il cibo, la qualità, il territorio, la passione del territorio e il *genius loci* sono tutte questioni che creano una ricchezza che va ben oltre il fatturato del Prosecco, ma insieme ad altre componenti creano esattamente quella ricchezza, quella produzione e quel *brand* Italia che consentono al nostro Paese di essere un punto di riferimento a livello mondiale. I dati che molti colleghi hanno fornito in realtà riguardano solo uno dei tre consorzi, il Prosecco DOC, perché dovremmo poi aggiungere anche gli altri: quello di Conegliano Valdobbiadene e quello di Asolo. La produzione di bottiglie è ormai di più di 600 milioni all'anno e

C'è da dire che i produttori, tra l'altro, anche con difficoltà, hanno rimodulato i canali di vendita: è esploso anche l'*e-commerce*, di cui nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 325 in Giappone c'è stata una crescita del 224 per cento; c'è davvero quella genialità capace di lavorare non solo il prodotto, ma anche il processo e la comunicazione, che sono i tre elementi centrali che fanno

Cosa potrebbe essere dello Château Lafite o dello Champagne? Cosa potrebbe essere dei vini tradizionali, se si apre la porta a una deriva di questo tipo? Dove vanno la qualità e la tutela dei consumatori, come diceva giustamente il senatore Taricco? Dove va la credibilità dei prodotti, soprattutto italiani, ma anche a livello europeo, dove pure ci sono delle eccellenze? Signor Ministro, la invitiamo davvero a fare squadra con Francia, Spagna e tutti i Paesi che hanno tutto l'interesse a combattere insieme.

a portare una riflessione e a fare anche una grande battaglia in questo senso all'interno dell'Unione europea, non solo genericamente sulle denominazioni,

Non è un caso, tra l'altro, che il valore di quel territorio sia stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha iscritto le colline del Prosecco del Prosecco nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Questo è l'altro elemento. Queste due questioni, la difesa della denominazione del marchio e quella del territorio, sono assolutamente e strettamente legate. Si tratta della

Credo che il dato più importante, da questo punto di vista e dal punto di vista giuridico, sia stata proprio la sentenza della Corte di giustizia europea - che lei ha citato poco fa,

Il regolamento europeo protegge le produzioni DOP da condotte relative sia ai prodotti sia ai servizi; non può quindi esistere, nel

del centro di Roma. innanzitutto la non omologazione, in un'epoca di globalizzazione di tutto quello che mangiamo, di come ci vestiamo e spesso anche di come pensiamo. Credo che questo sia un elemento assolutamente fondamentale.

l'abbiamo vinta. Anche sul Prosecco oggi credo si stia lavorando: come sa, il pericolo della monocoltura è notevole; molti produttori, infatti, stanno diventando anche la punta di diamante di un processo che punta in modo spasmodico sulla qualità

l'idea di un modello agricolo e produttivo e di una qualità dei prodotti che non possono trovarsi dovunque, ma che hanno un legame profondo con una

per portare avanti questa battaglia contro l'ennesima appropriazione indebita dei nostri marchi.

con poco stupore, a parer mio, questo è l'anno del Prosecco. Si è raggiunto un totale di 600 milioni di bottiglie prodotte in nove province del Nord-Est italiano, che vanta tre denominazioni d'origine. un vero e proprio universo enologico, che durante i mesi pandemici si è distinto per filiera fatta bene e innovazione; ha resistito allo *shock* dei mercati e ha addirittura incrementato le vendite, aprendosi a nuovi canali come *e-commerce* o *app*. *boom* anche per il Prosecco rosé, che con 37 milioni di bottiglie vendute in sei mesi si conferma prodotto d'eccellenza, amato soprattutto negli Stati Uniti e in Germania, Regno Unito ed Estremo Oriente. questa non è solo resilienza, ma capacità imprenditoriale, pragmatismo e lungimiranza, che rendono il solo e unico Prosecco un prodotto inimitabile e richiestissimo a livello mondiale. Come accade per tantissimi prodotti italiani, però, gli introiti derivanti da *business* fanno gola a tanti. Questa è la volta della Croazia, che ci prova. In questa settimana discutiamo infatti della possibilità di riconoscimento del *Prošek* croato.

è il fatto di ritrovarci ancora una volta in quest'Aula a lamentare ciò che potrebbe essere un pericoloso precedente a danno del *made in Italy*. C'è chi pensa che non esistano rischi di confusione tra Prosecco e *Prošek*. Non penso sia così. Semmai, non esistono rischi di confusione per gli intenditori di Prosecco, ma pensate a un consumatore che si affaccia per la prima volta sulla miriade di vini in commercio: abituato probabilmente al vino che generalmente in Italia, come direbbero le nonne, si usa in cucina, ma con il quale non si brinda, quale non si brinda, avendo spesso sentito parlare di Prosecco, decide di andare al supermercato e provare il *Prošek*, più economico e dal nome quasi simile. Si ritroverà a bere un vino fermo e non proverà l'esperienza delle nostre pregiate bollicine, che da sempre accompagnano i momenti belli e da ricordare; di fatto, berrà un passito dolce, che nulla ha a che fare con le caratteristiche secche del nostro Prosecco italiano; per lui quello sarà semplicemente Prosecco, indipendentemente dal fatto che alla fine apprezzerà o no il prodotto. Il ragionamento, però, indigna ancora di più perché porterebbe ingenti danni per i nostri produttori che guidano le esportazioni. Non credo di sbagliare quando dico che, se la richiesta croata dovesse essere accolta, ci troveremmo di fronte, come hanno detto già i miei colleghi, a un vero e proprio fenomeno di *italian sounding* legalizzato dall'Europa. Tutto ciò sarebbe inaccettabile, visto e considerato che l'*italian sounding* genera un giro di *business* ai danni dei produttori italiani da 100 miliardi l'anno. Cosa accadrà dopo il *Prošek*? Daremo man forte a prodotti come il Parmsan o la salsa Pomarola? Assolutamente no: ecco perché il *Prošek* è un precedente da evitare. Cosa c'è da fare? Sicuramente continuare a parlarne, signor Ministro: il dibattito non deve mai affievolirsi. Inoltre, in sede europea bisogna presentare un ricorso completo di tutte le nostre obiezioni motivate, al fine di far comprendere alla Commissione come dietro alla semplicità di un nome ruotino reputazioni e introiti di un settore traino del PIL italiano. È altresì fondamentale cercare di far capire che, quando si parla di prodotti italiani, non bisogna farlo con leggerezza; bisogna piuttosto agire su un fronte comune a livello europeo, al fine di tutelare un comparto, quello dell'agroalimentare italiano, che anche durante la pandemia ha permesso di portare sulle tavole di tutti i cittadini europei, e non solo, prodotti di eccellenza e con altissimi *standard* qualitativi. Per questo siamo sempre grati ai nostri imprenditori. Forza Italia c'è, è al fianco suo e degli imprenditori.

di questa iniziativa della Croazia che, tramite la Comunità europea, sembra voler registrare la denominazione del Pro*š*ek.

11.500 aziende che lavorano tutte nel settore del Prosecco in 23.000 ettari, con una superficie media di due ettari per ogni azienda; abbiamo giovani che lavorano in questo settore ed è una cosa molto piacevole e innovativa avere giovani che si riavvicinano alla terra e che credono nel futuro del loro territorio.

ha permesso agli agricoltori anche di risollevarsi economicamente, oltre a essere un'eccellenza del *made in Italy*. I numeri del prosecco sono eccezionali ne abbiamo visto una continua crescita. I numeri del Prosecco ci permettono - me

a nome di tutti i colleghi, perché veramente si conferma che siamo sul pezzo - siano state riconosciute patrimonio dell'UNESCO. C'era l'allora ministro e oggi sottosegretario Centinaio; c'era il nostro governatore Luca Zaia, che e si è impegnato moltissimo per il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'UNESCO. tratti sicuramente di un fiore all'occhiello dell'italianità nel mondo. L'UNESCO riconosce le nostre colline patrimonio dell'umanità, alla fine questa è la sostanza, ma poi vediamo che la Commissione europea

Ministro, sta nel fatto che, se passa la dicitura Prošek, apriamo un foro nella diga, quella che oggi sta proteggendo tutto l'*italian sounding* ed è a salvaguardia di tutti i prodotti

che diventerà visiva nel momento in cui si produrranno delle bottiglie, come ci ha fatto vedere il presidente Vallardi. Questo è certamente un grande pericolo per la nostra economia. L'Italia

Così come sarà fondamentale e di fondamentale ausilio l'attivazione del tavolo tecnico per sostenere i produttori italiani del Prosecco nel ricorso contro la Commissione UE. Ovviamente quando si elaborano dei documenti, chi fa da sé non fa granché in realtà, come mi è stato insegnato in questo caso il Ministero realizzerà il tavolo tecnico attraverso chi lavora all'interno del settore e del comparto, quindi i consorzi. assurdo pensare che seppur nella fase istruttoria dell'intera procedura di registrazione in Europa del Prošek, la Commissione UE abbia comunque concesso il primo sì verso quella che è a tutti gli effetti la violazione del divieto di utilizzare nomi che

È proprio così, trattasi di un vero e proprio raggiro nei confronti dei consumatori, i quali, al momento dell'acquisto, nonostante i prodotti siano di diversa qualità, vengono fuorviati dall'omonimia della denominazione utilizzata e dalla somiglianza che ne deriva. La vicenda di cui si discute dimostra come il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo, venga spesso intaccato. Di certo non possiamo permetterci di non difendere le nostre preziosità di fronte ai vari e non rari attacchi da parte di coloro che nei fatti attuano vere e proprie pratiche di concorrenza sleale. Questo è: concorrenza sleale. Anche perché occorre considerare come per la produzione dei vini DOP e ad indicazione geografica tutta una serie di requisiti, i quali vengono nel tempo rivisti in chiave sempre più stringente. Viene pertanto richiesto un legame sempre più forte con il territorio da cui provengono, di cui siamo stati proprio noi vittime, come prima si si è detto più volte relativamente al Tocai friulano, perché aveva una denominazione troppo simile al Tokaji ungherese e slovacco e abbiamo dovuto noi fare un passo indietro con il nostro nome. Adesso invece dobbiamo fare cinque passi avanti e chi sta attuando questa pratica scorretta ne deve fare Ci si aspetta quindi che dinanzi a tali condizioni richieste circa la natura, la qualità e la vera origine del prodotto, non si possano poi ammettere pratiche scorrette come un tale caso di omonimia. sarebbe un grande controsenso, chiaro e visibile a tutti. In conclusione, una denominazione storica come quella rappresentata dal Prosecco DOC e dal Prosecco con così come tutte le denominazioni europee e le eccellenze protette, va tutelata unitamente alla garanzia per il consumatore e alla tutela del territorio e delle tradizioni. Resto pertanto fiducioso anche io, come il Ministro, circa il lieto fine di questa assurda vicenda. Grazie, Ministro, per quello che sta facendo.

Grazie,

sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Dichiaro aperta la discussione generale.

In ogni caso, signor Presidente, la riforma risponde esattamente al concetto di giustizia penale che ha questo Governo, che

i colletti bianchi, i politici, gli amministratori, i ricchi insomma devono essere tutelati e devono avere ampie possibilità di immunità. La riforma

estendendo il patteggiamento, ampliandone (a favore del reo naturalmente) gli effetti alle pene accessorie, alla confisca, agli effetti extrapenali della sentenza. Inoltre, ad esempio, estende l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Elencherò, signor Presidente, qualcuno di questi reati che adesso potranno non essere puniti se particolarmente tenui. Mi dica lei se possono essere tenui l'istigazione alla corruzione, la falsa testimonianza, l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'agevolazione alle comunicazioni dei detenuti al 41-*bis*, l'inquinamento ambientale, il traffico illecito di rifiuti, la falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, lo sfruttamento del lavoro, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'usura e l'autoriciclaggio. Tutti questi sono reati che sono puniti con una pena non superiore, nel minimo, a due anni. Ovviamente, il massimo è molto più alto, ma vi è l'*escamotage* di cambiare. Prima,

nella rete, potranno essere dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto. Avete sentito bene quali sono i tipi di reati di cui stiamo parlando. Ancora, si estende l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento. Vieni prosciolto in primo grado? Il pubblico ministero non può fare appello. Ancora, viene estesa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato per pene fino a sei anni.

deterrenza del codice penale rispetto a coloro che potrebbero pensarci due volte prima di commettere dei reati e che sapranno perfettamente che potranno farla franca. Il carcere è previsto, sostanzialmente, soltanto per i poveracci. Il capolavoro, in questo senso, è proprio l'improcedibilità per il superamento del termine di durata dell'appello o del ricorso in Cassazione. È vero che vengono previste delle possibilità di proroghe,

bisognerà dimostrare che è particolarmente complesso. E su quella motivazione e su quel provvedimento potrà essere fatto ricorso in Cassazione. Quindi, è facile immaginare che, per tutti i reati, compresi quelli di mafia, dove vi è la possibilità di proroga e deve esserci sempre questa motivazione, rei, che sono stati anche condannati in primo grado, faranno sicuramente ricorso. E in Cassazione si discuterà non se siano colpevoli o innocenti, ma se la motivazione per chiedere la proroga è stata corretta, puntuale e avrà dimostrato che c'era una particolare complessità.

è la seguente: le procure vengono sottoposte alle indicazioni della politica al fine di graduare i reati che dovranno essere perseguiti. È evidente il concetto. Il concetto è che,

un potere del tutto autonomo. Si vogliono ridurre a un fascio tutti i poteri; a un fascio tutti i cittadini. Il Parlamento deve essere allineato, i partiti devono essere allineati. Che cosa vi ricorda questo? Chi è che Chi è che ha preso ispirazione dal concetto che tutti devono essere allineati come dei fasci stretti in una fascina? Signor Presidente, a questo punto devo dire due parole anche su come si è svolta questa discussione. Stiamo parlando di una riforma che avrà delle conseguenze disastrose nella pratica, ma ancora più disastrose dal punto di vista del segnale che viene dato alla società, dal punto di vista culturale. Ripeto, infatti, che qui la volontà è proprio quella, in tutti i tasselli, di dire: il Governo detta, il Parlamento esegue. E che cosa detta il Governo? Detta esattamente questo: due velocità, due tipi di giustizia. Per i ricchi e per i potenti, immunità

perché in Commissione ieri è arrivato il momento di parlare degli emendamenti e immediatamente, il giorno stesso,

Ieri non abbiamo votato un solo emendamento: è questo il concetto che avete del Parlamento? E lei, Presidente, non fa nulla per difenderlo? Stiamo dando un esempio che in futuro verrà ricordato. Questa è una tragica pagliacciata e siccome questo Parlamento sta diventando un circo che schiaccia soltanto i pulsanti, non esistono pagliacci e circhi senza i palloncini.

Senatore Crucioli, la invito ad agevolare l'intervento degli assistenti, altrimenti questo diventa un richiamo formale, con tutte le conseguenze del caso.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

Presidente,

che non sono calate dall'alto, ma sono impegni precisi che ha assunto il nostro Paese con riferimento agli atti relativi al programma di Governo e quindi anche al *recovery* *fund.* L'intervento che ho ascoltato prima mi induce a fare una piccola valutazione, perché ho ben chiaro in mente

democrazia parlamentare da chi progettò quel tipo di normativa, assumendo degli impegni che poi vennero disattesi. *(Applausi)*. Questo lo devo dire.

può capire bene quale sia la mole del lavoro svolto, soprattutto al di là delle ultime mediazioni relative alle improcedibilità per la costruzione di un testo

contrario. Abbiamo avviato la legislatura con una conflittualità altissima su questi temi; è proseguita una conflittualità altissima, oggi, invece, siamo qui a discutere di un punto di equilibrio, che può soddisfare o meno. Forza Italia lo ha detto anche durante il dibattito alla Camera negli interventi che si sono susseguiti: avrebbe preferito qualche norma in più, e però, indipendentemente da questo, si è assunta la responsabilità di trovare un testo condiviso.

fa scalpore sui giornali e, senza aver avuto di fatto neanche uno straccio di sentenza di primo grado, si trova rovinato da un processo mediatico e nessuno lo può ripagare. Abbiamo visto sfilate di politici che sono stati assolti dopo aver avuto reputazione, carriera e famiglia

Si è parlato molto di una serie di temi, che però lascio a chi, magari, ha una cultura da penalista più attenta; io vorrei ricordare l'importanza di questa riforma con riferimento ad altri aspetti di cui forse si è parlato meno. È una legge delega che contiene una serie di indicazioni precise, ad esempio, in riferimento al processo penale telematico e al malfunzionamento dello stesso. Vorrei ricordare che i penalisti e le camere penali tante volte sono intervenuti su questo tema, perché un processo che sia ben fatto, ai giorni d'oggi non può prescindere da tutte quelle misure che riguardano la digitalizzazione, che velocizzano e semplificano di per sé le procedure. Questa delega è completa da questo punto di vista e prende in esame i vari aspetti che devono essere messi in evidenza.

alla famosa udienza, che oggi è diventata solo un'udienza filtro relativa al rinvio a giudizio, che doveva servire a mettere dei punti con riferimento all'andamento del processo. Oggi, con il principio della ragionevole previsione della condanna, si torna a quell'orientamento perché sia attuato, non perché ci si trovi di fronte semplicemente a un passacarte, per intenderci, o a un copia-incolla, bensì a un'analisi più seria su cui basare la volontà di rinviare o meno a giudizio una persona.

che magari, tolta di mezzo la conflittualità in particolare tra Forza Italia e la magistratura, si sarebbe risolto tutto. Invece questa legislatura ha dimostrato esattamente l'opposto: la conflittualità è stata altissima e, per certi aspetti, possiamo tranquillamente dire che

piazza, per dare gioia a chi viene a vedere il rogo, ma è una persona che dallo Stato deve avere un processo giusto, equo, razionale e, soprattutto, di ragionevole durata. Questo per me è stato un momento di importante svolta e mi auguro che il Paese, che ha finalmente la possibilità di instradarsi su questa strada, che è quantomeno razionale e posta nell'alveo nella Costituzione, non la abbandoni

mi auguro, per me stessa, per voi tutti e per le generazioni a venire, sia terminata o comunque stia per terminare.

nel dibattito politico sentiamo spesso dire che la finalità principale della legge delega per la riforma del processo penale è quella di rispondere a un'esplicita richiesta, rivolta all'Italia da parte dell'Unione europea, ossia quella di risolvere il fondamentale problema dell'eccessiva durata dei giudizi, che poi sappiamo si risolve sempre in denegata giustizia, e ciò al fine di rendere il Paese più appetibile agli investitori e favorire così la ripresa economica. In realtà questa è una riforma che ci chiedono prima di tutto i cittadini, i cittadini, che ormai da vent'anni assistono ad un lento declino del sistema giustizia, svuotato di ogni risorsa e al collasso, con processi troppo lenti numerosi, come provano le 1.202 condanne inflitte ad oggi all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la violazione del principio della ragionevole durata del processo. Le lungaggini sono sempre un gravissimo danno per la vittima, che ha legittimamente diritto al risarcimento, ma anche per l'imputato, che non può essere assolto dopo venti o trenta anni, ma - attenzione! - neanche condannato, essendo ipotizzabile che, in un ampio arco di tempo, vi sia stato un cambiamento della sua personalità. Ecco allora che con il Governo precedente, il Conte II, ma anche con l'attuale abbiamo cercato di risolvere il malfunzionamento del sistema giustizia sul lato penale, anche in questo caso con un enorme piano di assunzioni ordinarie, per circa 21 milioni, a cui si aggiungono quelle straordinarie, per 18 milioni. Ma le risorse non bastano per riformare la giustizia. Occorre anche un nuovo modo di intendere l'organizzazione degli uffici giudiziari e la stessa giustizia: non più tutto il carico di lavoro sul singolo magistrato o sul collegio, ma sullo staff del magistrato, con l'istituzione dell'ufficio del processo. Il magistrato non lavora più da solo, ma si avvale del contributo di diverse professionalità,

Questa legge delega ha previsto anche una disciplina organica del nuovo istituto della giustizia riparativa: un nuovo e concreto modo di concepire una risposta alla giustizia, nell'interesse della vittima e del reo, un vero e proprio atto di civiltà sociale e giuridica. È prevista nella legge delega la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e persino durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità. Abbiamo previsto anche un nuovo concetto di familiare della vittima, che da oggi non sarà più solo il coniuge, ma anche la parte di un'unione civile, civile, i parenti in linea retta (i fratelli e le sorelle) e le persone a carico della vittima. A questo proposito vorrei ricordare anche un ordine del giorno a mia prima firma, recepito da tutta la Commissione proprio ieri sera, affinché tutti i programmi di giustizia riparativa siano gratuiti. Riguardo invece all'esigenza di accelerare il processo penale, la legge delega prevede un rafforzamento dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato), al fine di renderli sempre più appetibili, con un effetto deflattivo sul rito dibattimentale.

amplia inoltre l'ambito di applicazione della querela, per i reati puniti con pena non superiore a due anni, e si potenziano gli istituti della non punibilità, come per la tenuità del fatto, nonché la messa alla prova;

A questo proposito, vorrei ricordare anche un'altra norma inserita - finalmente - nella riforma, quella dell'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati

una norma fondamentale per fermare tutti quei reati che precedono il femminicidio. Abbiamo pensato poi di estendere la portata applicativa del codice rosso anche alle vittime dei reati di violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio (quindi appunto il femminicidio). La legge delega di riforma del processo penale incide inoltre sulla fase delle indagini preliminari, anche qui subordinando l'esercizio dell'azione penale a criteri di priorità trasparenti e predeterminati, che saranno individuati con legge del Parlamento. Si tratta di una norma che, tra l'altro, avevamo già previsto nel codice rosso; la legge si chiama proprio codice rosso, perché prevedeva una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica. Un'altra novità molto importante è il ricorso straordinario alla Corte di cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: un mezzo di impugnazione nuovo, che va però a colmare una lacuna italiana di oltre vent'anni.

pesantemente con la collaborazione delle altre forze politiche per introdurre dei correttivi. Oggi, pertanto, i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati dal giudice in qualsiasi procedimento penale in presenza dei seguenti requisiti: complessità per numero di parti delle imputazioni; numero e complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare. Inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria, ossia le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire da gennaio 2020. Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente tre anni per l'appello e un anno e mezzo per la Cassazione. Soprattutto abbiamo preteso - siamo riusciti a introdurle - alcune proroghe per quanto riguarda i reati particolarmente gravi quali i reati per finalità di terrorismo e di eversione, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti. In questi casi il termine può essere prorogato senza limiti di tempo. Per i delitti aggravati con metodo mafioso si può arrivare a una durata massima dell'appello a cinque anni e per la Cassazione a due anni e sei mesi. I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano invece nei procedimenti puniti con l'ergastolo, anche con effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti e quando l'imputato vi rinunci. l'imputato vi rinunci. Presidente, questo è un nuovo modo di intendere il processo penale. È un modo che impone un cambio di passo per tutti i soggetti che ne sono protagonisti (magistratura e avvocatura), che sicuramente in alcune parti del territorio funzionerà, ma che in altre potrebbe anche lasciare delle sacche di impunità. Se questo sarà, occorrerà immediatamente un nuovo intervento legislativo che ne corregga le disfunzioni e a ciò saremo pronti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, oggi siamo a discutere una riforma del processo penale

Purtroppo c'è stato in questo periodo uno stravolgimento del progetto politico che aveva avuto il mandato popolare in favore di un progetto ormai

sappiamo bene aver operato anche nell'ambito della difesa dell'*ex* presidente Silvio Berlusconi. È stata partorita una riforma che stravolge il meccanismo costituzionale della giustizia penale

denaro, risorse ed energie per poter garantire la tenuta del patto sociale e lo stato di diritto in una sorta di azienda di disbrigo pratiche. pratiche. A questo è ridotta quella che una volta doveva essere la giustizia penale: una sorta di agenzia di disbrigo pratiche. Questa riforma viene varata con grande velocità, con dei passaggi a tappe forzate nei due rami del Parlamento, quindi sia alla Camera

del *diktat* del Governo, per arrivare a un approdo definitivo in tempi rapidissimi, col pretesto del collegamento della riforma con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento non si è potuto esprimere chiaramente né in in un ramo né nell'altro, con tutta la dovizia di confronto e di discussione che sarebbe stata indispensabile per partorire una riforma che garantisse veramente giustizia a tutti i cittadini, e non soltanto mettendo in campo delle strategie per garantire l'impunità

del primo grado di giudizio, che è stata introdotta per accontentare il MoVimento 5 Stelle, che doveva in qualche modo esibire un risultato di fronte ai suoi accoliti, dovendo giustificare l'adesione a questo Governo e, quindi, la partecipazione di alcuni Ministri all'interno delle compagine dell'Esecutivo. Ma in realtà è stato introdotto un istituto ancora più perverso, quello dell'improcedibilità, dell'improcedibilità, che mette una tagliola ai processi penali in secondo grado e in Cassazione, in funzione delle tempistiche di svolgimento dei due gradi di giudizio: due anni in appello, un anno in Cassazione. Eventuali richieste di proroghe, che comunque non possono superare i due anni, possono essere richieste solamente attraverso vie giurisdizionali. Quindi i processi, anziché abbreviarsi, si allungano perché si arricchiscono sempre di nuove richieste di proroghe e rinvii, di proroghe e rinvii, e si incentivano gli imputati, che sanno benissimo di non poter far valere efficacemente le loro ragioni attraverso le sedi giudiziarie, giudiziarie, a ricorrere in tutti i gradi di giudizio e ai riti ordinari, perché solo quelli possono garantire la cosiddetta tagliola, cioè che il processo a un certo punto decada e quindi non resti più traccia del reato (quando la Costituzione impone l'obbligo dell'azione penale), e non resti nemmeno più traccia sulla fedina penale. Pensiamo - ad esempio - a quanti politici sarebbero stati colpiti dalla legge Severino e avrebbero dovuto interrompere le loro brillanti carriere, portate avanti a discapito della collettività. Questa è la vostra bellissima riforma, che è contro l'interesse collettivo; una riforma che non dà giustizia, ma la nega; una riforma che, con il pretesto di efficientare

Avete negato la possibilità ai cittadini italiani comuni di avere una giustizia penale. Avete negato la possibilità alle vittime di vedere celebrata la giustizia per eventuali torti e danni subiti. Avete tolto fiducia nello Stato di diritto, perché ormai siamo tutti convinti di non vivere in uno Stato di diritto. Avete rotto il patto sociale che lega la società, per cui tenere una condotta eticamente e legalmente valida è ormai obbligatorio solo per chi non ha poi gli strumenti per difendersi nelle sedi di giudizio a ciò deputate, facendo valere i propri diritti di cittadino. Avete quindi ridotto i diritti di cittadinanza a tutti i livelli e vi siete procacciati un'immunità permanente, oltre ad averla garantita garantita con lo scudo penale a tutti coloro che oggi praticamente, su vostra delega, stanno agendo, discriminando le persone, abusando del loro ruolo per compiere atti nefasti e criminali. State quindi praticamente tutelando un sistema che si gestisce a uso e consumo

giustizia. Naturalmente dire che c'è una discussione è un'affermazione grossa perché, mentre in questo momento i capi politici - vedo che anche l'Aula del Senato è mezza vuota

qui in Parlamento, nelle Aule del Parlamento italiano, organo al quale la Costituzione attribuisce la funzione legislativa, si sta uccidendo la democrazia.

e viene impedita anche oggi, perché sappiamo che il Governo su questa riforma porrà per ben tre volte la fiducia. volte la fiducia. Bisognerebbe fermare questa riforma, che non migliorerà la giustizia italiana, ma la comprometterà. Che la prevista riorganizzazione del diritto penale presenti più ombre che luci non lo dico io, anche se umilmente avrei qualche competenza per farlo. Lo dicono autorevoli magistrati e operatori che sono in prima linea, in trincea tutti i giorni a combattere la criminalità organizzata e tutto il malaffare presenti in Italia. Al di là di ogni polemica politica, bisogna ragionare su dati oggettivi. Non è un caso che a lanciare l'allarme siano

chiunque. Nel corso di una recente intervista Nicola Gratteri, procuratore antimafia, ha commentato la riforma Cartabia in modo diretto e senza fronzoli, dicendo chiaramente che è la peggiore riforma da quando è in magistratura e definendola devastante e dannosa. Si tratta di due termini che onestamente fanno tremare le vene.

Matteo dice che l'approvazione della riforma con il meccanismo della improcedibilità per decorso del tempo in appello e Cassazione rischia di segnare una grave sconfitta per la giustizia, che la riforma rischia addirittura di rafforzare i poteri criminali che da sempre si pongono come regolatore di conflitti della società. A poco o nulla valgono la distinzione che la ministra Cartabia fa tra una Corte d'appello e un'altra, oppure la trovata - aberrante, dal mio punto di vista - di creare una Commissione giustizia al Sud,

si sta facendo un passo indietro. Abbiamo votato cantando la riforma Bonafede, che pure era un segnale forte che abbiamo dato. dato. Ora, per coerenza, non dovremmo tornare sui nostri passi, ma lo stiamo facendo. Invece di confermare e perfezionare una riforma della giustizia quella di Bonafede, che pure era stata avviata - si stanno distruggendo tutto il lavoro fatto in questi anni e anche gli importanti risultati raggiunti

La speranza è che questo andazzo finisca presto e il Parlamento torni ad essere il luogo di confronto e democrazia dove si promuove, si discute, si dibatte e si corregge per raggiungere poi decisioni politiche e sostanziali - ho una visione molto laica della politica: la politica è servizio per il benessere dei cittadini e della Nazione - e non resti un luogo dove si continuano a ratificare decisioni. Mi rivolgo a tutti i colleghi di buon senso in quest'Aula: possiamo ancora fermarci. Fermiamo questa devastante riforma del diritto penale. È stato anche detto che non ce lo chiede l'Europa, che ci ha chiesto

Questo è evidentemente quello che sarà il Parlamento che qualcuno vuole, introducendo attraverso le firme digitali la democrazia diretta, tanto cara del MoVimento 5 Stelle, che - per carità - ha una sua filosofia sulla quale ho qualche perplessità. Evidentemente però una ragione indiretta c'è nel ritenere che questi avrebbero anche ragione, visto che qui non c'è nessuno a discutere della riforma del processo penale. Credo che la Presidenza del Senato dovrebbe fare un rilievo a tutti i parlamentari. C'è questione e questione e la questione afferente alla riforma del processo penale interessa tutti i cittadini. Entrando nel merito,

il cosiddetto fine processo mai. Si ristabilisce il diritto sostanziale e lo si fa utilizzando un orologio ordinario e un orologio sulla sfera di Greenwich consentitemi l'espressione - e cioè la prescrizione del reato e la prescrizione del processo che attiene all'improcedibilità, secondo di nuovo conio, sul quale sicuramente ci saranno anche dei problemi di valutazione e di inferenza rispetto al diritto sostanziale e al diritto processuale. Credo che la materia della prescrizione sia materia ampiamente consolidata nella giurisprudenza e quindi

che scandisce la vita di ognuno di noi e rende di per sé irrilevante ricercare una punibilità, ad eccezione dei reati più gravi, viene ristabilito con questa legge delega. quindi grande apprezzamento per il lavoro che è stato fatto. Tuttavia, devo anche precisare che forse non ho colto alcuni aspetti

il fatto che viene sottaciuto - ed è pericolosissimo - l'inserimento della pesca a strascico attraverso i *trojan,* attraverso i captatori informatici, anche per i reati che non hanno nulla a che fare con quelli più violenti, i reati di mafia, che sono fondati sulla violenza, bensì per i reati contro la pubblica amministrazione. L'uso improprio del fotocopiatore, che si chiama peculato, può essere oggetto di intercettazione *trojan* anche al di fuori dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Vogliamo mettere fine a tutto ciò?

e ha ridicolizzato il Parlamento, non sapendo però che ridicolizzava anche sé stesso. Perché non è qui ora? Dovrebbe essere qui ora, perché chi rivendica la mancanza di dibattito è il primo che, terminato il suo intervento, se ne va. E, quindi, non può dire che è stato un attentato alla democrazia.

per cortesia: si è appena richiamato alla dignità del Parlamento, sia conseguente.

tutela la segretezza delle comunicazioni con una riserva di legge e con una riserva di giurisdizione: tutte queste cose le abbiamo perse. Io invito il Governo a riflettere

ma risolvere delle questioni che erano aperte, per esempio gli effetti extrapenali del patteggiamento. In tale caso, con questo provvedimento si fa chiarezza su questi aspetti. Si introduce un allargamento dei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. E si interviene nell'appello, introducendo dei filtri reali e soprattutto un principio fondamentale, che ha visto Forza Italia quale prima forza politica ad affermare con la legge Pecorella, di cui noi rivendichiamo bontà e la finalità, il principio della non appellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado con formula piena. *(Applausi)*. Qui si introduce finalmente la possibilità per il legislatore, in questo caso per il Governo attraverso il decreto legislativo, di introdurre la non appellabilità della sentenza della sentenza di proscioglimento per i reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa pecuniaria. È già qualcosa; è già un prendere atto che quelle sentenze della Corte costituzionale, che chiaramente risentivano di un principio, sono state superate.

come diceva stamattina la collega Modena, della quale non posso che condividere l'augurio

Presidente, sono evidentemente delle situazioni così gravi e dei torti così profondi che giammai potranno essere risarciti.

stiamo discutendo di una riforma che possiamo definire epocale.

può solo ossequiosamente approvare le norme scritte dall'Esecutivo, senza alcuna possibilità di esercitare le funzioni che gli sono riconosciute dalla Costituzione e che vengono esercitate in nome del popolo e dei cittadini. Il provvedimento è arrivato blindato alla Camera e qui al Senato la Commissione giustizia non ha avuto il tempo di esaminare i numerosissimi emendamenti presentati dai parlamentari: nessun confronto, nessuna possibilità di modificare il testo, nessuna democrazia. E questa volta non ci sono le esigenze di necessità e urgenza che hanno giustificato, negli ultimi mesi, le limitazioni al dibattito parlamentare. Non siamo di fronte ad un decreto-legge, ma ad un disegno di legge che vuole riformare il processo penale, una materia che a che fare con le libertà fondamentali e che richiede più che mai ponderazione e confronto. La riforma Cartabia incide su principi fondamentali del processo penale: il principio di oralità e di obbligatorietà dell'azione penale. Questa riforma presenta criticità gravissime, almeno per quanto mi riguarda (poi siamo in Parlamento e ognuno ha le proprie opinioni), e sono proprio gli addetti ai lavori, i magistrati, a dirlo; a partire da Gratteri, che ha dichiarato che questa è la peggiore riforma di tutte e che se fossero in vita Falcone e Borsellino salterebbero dalla sedia leggendo il termine improcedibilità. Nino Di Matteo ha parlato di «mortificazione dei diritti delle parti offese» e di un «diffuso senso di sfiducia dei cittadini verso la giustizia». Anche la mia collega Granato ne ha parlato e ha fatto degli esempi qualche minuto fa. Ritengo che questa riforma voglia risolvere i problemi della giustizia legittimando le attuali carenze del sistema. I processi sono lunghi? Benissimo, li eliminiamo. Non ci sono gli strumenti necessari per garantire i diritti degli imputati? Eliminiamo i diritti, ovviamente. A queste criticità Sinistra Italiana ha tentato di porre rimedio rimedio attraverso approfondite elaborazioni e numerosi emendamenti, presentati da me e dalle colleghe Doriana Sarli, Paola Nugnes ed Elena Fattori, oltre ad un ordine del giorno, presentato sia alla Camera che al Senato, che impegnava il Governo ad assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo per il reato di disastro ambientale, introdotto nel 2015 e previsto dall'articolo 452-*quater* del codice penale. Infatti, con questa riforma della giustizia i criminali che avvelenano l'ambiente non saranno puniti. Una criticità inammissibile, che rischia di rendere vani i seppur pochi passi in avanti fatti finora dalla normativa relativa al disastro ambientale. Infatti, tra i reati gravi per cui è consentita la proroga mancano i reati ambientali, che - come la storia italiana dimostra - necessitano di processi giudiziari lunghi e molto complessi. La riforma Cartabia rischia di regalare l'impunità a chi distrugge i territori avvelenando chi li abita. *(Applausi)*. Va infatti ricordato che l'inquinamento ambientale non si ferma con la via del processo, come avviene ad esempio con i delitti. Una persona la uccidi una volta, l'ambiente lo uccidi ogni giorno. Quindi, non sono reati circoscritti nel tempo ed è giusto non fissare limiti di tempo per i relativi processi. Come non pensare al disastro del fiume Sarno o della terra dei fuochi? Com'è possibile regalare l'impunità ai criminali che hanno avvelenato la Campania, la mia terra, e ucciso migliaia di persone? gli emendamenti che ho presentato affrontavo numerose criticità. Innanzitutto, la riforma Cartabia prevede che sia il Parlamento, con una legge, a stabilire le modalità generali in virtù delle quali le procure della Repubblica dovranno indicare i criteri con cui dare priorità alle notizie di reato, da trattare quindi con precedenza rispetto alle altre. Questo confligge con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e, come denunciano i magistrati, rischia di violare l'assetto costituzionale. Inoltre, si prevede che i decreti legislativi per la riforma del processo siano adottati di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e acquisito il parere della Conferenza unificata e ciò è incomprensibile: vista la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, cosa c'entrano le Regioni in questa fase decisionale? Un'ulteriore criticità è relativa al fatto che il testo delle riforme prevede che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite direttamente dal difensore. Ma perché mai gli avvocati dovrebbero mettersi sulle tracce dei propri assistiti, sostituendosi allo Stato? La riforma prevede la registrazione audiovisiva come ulteriore forma di documentazione dell'interrogatorio solo qualora gli uffici dispongano dei mezzi tecnici, quindi dei registratori. Sarebbe invece importante, a garanzia di chi viene sentito, che si procedesse alla registrazione audiovisiva sempre. È inaccettabile che in una riforma che vuole dare nuova vita al processo si faccia riferimento all'indisponibilità degli strumenti tecnici necessari e non si provveda invece ad acquistarli e ad incrementali. Ma dove siamo? È ugualmente inaccettabile prevedere che il ricorso all'appello, quindi il secondo grado di giudizio, sia inammissibile per mancanza di specificità dei motivi: così si viola il diritto dell'imputato di impugnare personalmente la decisione, costringendolo a tecnicismi che non appartengono al suo linguaggio e ledendo così i suoi diritti. Inoltre, Inoltre, uno degli emendamenti che ho depositato è mirato ad eliminare la previsione per cui davanti al massimo organo giurisdizionale, qual è la Corte di cassazione, non sia possibile partecipare all'udienza. L'oralità del processo è un principio irrinunciabile. Infine, ho proposto alcune modifiche atte ad intervenire sul sistema della prescrizione attualmente previsto dal testo, perché di fatto con questo provvedimento i processi evaporeranno, spariranno. Con i cavilli che contraddistinguono il sistema italiano, sarà possibile per gli avvocati cercare di far sforare i limiti stabiliti facendo sfumare così il processo e rendendo inutile il lavoro dei giudici di primo grado e del e ciò soprattutto per i processi più complessi e dunque più lunghi. Peggio di così questo Governo non poteva fare. Si legittimano le carenze esistenti, strutturandole in un sistema che cancella i processi più importanti e dando molte più opportunità ai criminali per farla franca.

signori del Governo, care colleghe e cari colleghi, desidero preliminarmente rivolgere, anche in questa circostanza, un ringraziamento

di doverlo fare anche verso il sottosegretario Sisto, che ha davvero dato un contributo fattivo, con un'opera di mediazione talvolta non facile, che a mio parere ha prodotto un ottimo risultato. Devo ringraziare anche i colleghi della Camera, che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Desidero iniziare questo mio intervento affermando prima di tutto il mio convinto appoggio a questa riforma, soprattutto perché segna la fine dello sfrenato giustizialismo che ha animato le riforme talvolta insensate degli ultimi anni. Abbiamo visto anche poco fa che c'è chi sostiene queste riforme senza poi probabilmente considerare il fatto che il nostro Paese ha bisogno di ben altro.

cavalcando il più delle volte - lo abbiamo visto anche poco fa - l'onda dell'emotività piuttosto che perseguire l'intento di dare al Paese un sistema in cui la giustizia sia anzitutto giusta ed equa. Si disegna quindi un sistema

quei diritti che - si badi bene - sono perfettamente delineati nella nostra Costituzione. Una delle cose che ho apprezzato maggiormente della ministra Cartabia è che fin dal primo giorno ha detto la Costituzione è stata e sarà sempre il faro di tutta la sua attività. Ebbene, forse tutti quanti dovremmo uniformarci a questo orientamento, a questo precetto. Tante volte ho giurato fedeltà alla Costituzione e credo fermamente in ciò che la ministra Cartabia ha detto: uniformiamoci alla Costituzione e sicuramente otterremo i risultati che questo Paese aspetta da noi. La riforma è sicuramente perfettibile, come tutte le leggi - l'ho detto molte volte in questi giorni - ma ottiene, tuttavia, un risultato straordinario che auspichiamo da sempre. Oggi, infatti, mettiamo finalmente fine all'attività che aveva caratterizzato il precedente Governo, che non ha esitato, per i motivi già detti più volte, a mortificare i diritti e le garanzie dell'individuo, finendo per mortificare, però, se stesso, e infatti ha dovuto cedere la mano al Governo Draghi affinché quei diritti venissero finalmente salvaguardati. Con questa riforma si attua quel concetto di processo penale che è stato mortificato troppe volte, secondo cui si ha un insieme di garanzie, che troviamo affermate nella Costituzione, per affrontare e decidere circa la violazione dei precetti posti a tutela della società e degli individui che la compongono, quindi del corretto svolgimento della vita sociale. in questa attività non si può prescindere dai valori che vanno dalla inviolabilità della libertà personale al principio di legalità fino ad arrivare all'autonomia della magistratura, al giusto processo e alla sua ragionevole durata. Oggi, quindi, compiamo un enorme passo avanti verso il processo giusto, che prima di tutto deve essere un processo agile e veloce, che possa avere una ragionevole durata così da andare anche a beneficio dell'imputato, sia esso colpevole o innocente. Badate, anche l'imputato colpevole è pur sempre un uomo, e come uomo che ha sbagliato, per i motivi più disparati, il suo percorso di vita, ha diritto a non aspettare tempi infiniti per l'accertamento dei fatti e per l'attuazione della risposta sanzionatoria, che deve essere pronta, immediata ed equa. E ciò anche per la riaffermazione di valore di quel comportamento che è stato punito e per avviare il processo di rieducazione che comunque deve improntare la risposta punitiva dello Stato. Solo in questo modo potremo rendere un servizio doveroso anche alle vittime dei reati, le cosiddette parti offese. Abbiamo sentito dire spesso che il processo che non si prescrive va a beneficio delle vittime: è una follia completa, una falsità. Le vittime vengono tutelate se il processo è veloce, non se abbiamo il fine processo mai, come inopinatamente aveva stabilito la riforma attuata dal Ministro della giustizia precedente, per essere chiari, quello che aveva che aveva le idee confuse sui concetti di dolo e di colpa. In questa direzione va la riforma che ci apprestiamo ad approvare. Si pensi all'avvio graduale del processo penale telematico o al sistema delle notificazioni, con la concentrazione dei tempi per gli avvisi e per le comunicazioni; all'incentivazione dei riti alternativi, rispetto ai quali - questo lo voglio sottolineare - forse avremmo potuto fare anche qualcosa in più; avremmo dovuto essere forse un po' più coraggiosi, rendendo più conveniente la decisione di non andare a dibattimento in più circostanze. Ovviamente avremmo ottenuto una riduzione più imponente dei carichi processuali e dibattimentali. Tuttavia, ciò che conta a mio avviso è che questo processo sia stato finalmente avviato, perché il resto potrà farsi cammin facendo. Da noi un vecchio proverbio dice - lo dico in italiano - che durante il percorso si aggiusta il carico, ed è questo che dovremo fare. Dovremo, cioè, apportare quelle piccole modifiche che si renderanno necessarie una volta che il nuovo sistema andrà a regime. Un altro aspetto che segna indubbiamente un cambio di passo rispetto all'impianto originario della riforma Bonafede è la questione della priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si sceglie infatti, finalmente, di affidare al Parlamento il compito di stabilire periodicamente i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si tratta di criteri generali, nell'ambito dei quali gli uffici del pubblico ministero saranno chiamati a individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei processi organizzativi. Affidare al Parlamento questo importante e delicato compito, visto l'enorme carico giudiziario, vuol dire garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, sottraendola all'esercizio discrezionale delle singole procure, che troppe volte hanno creato problemi nel sistema.

in tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, e il secondo prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Colleghi, questa per noi è davvero una priorità, perché si tratta di una previsione significativa e molto attesa, che garantisce maggior tutela e protezione alle vittime di maltrattamenti e di *stalking*

Devo sottolineare poi che importante e significativo è il ridimensionamento della prescrizione, anche se il "fine processo mai" è rimasto purtroppo per alcuni reati.

Quanti Enzo Tortora esistono nel nostro Paese? Quante persone innocenti vengono coinvolte con accuse infamanti, che poi vengono regolarmente a terminare nel nulla? Forse noi stessi e scusatemi se lo dico con uno sfogo...

stessi avremmo dovuto fare qualche riflessione in più, anche quando, in quest'Aula, abbiamo autorizzato l'arresto di un collega, che dopo cinque anni è stato dichiarato innocente perché il fatto non sussiste. *(Applausi)*. L'abbiamo messo in carcere:

per sottolineare che Italia Viva c'è su queste riforme, per dare una giustizia equa, giusta e soprattutto coerente con i principi costituzionali. Continueremo ad appoggiare la vostra azione, in questo senso e in questa direzione, che mi sembra davvero la più giusta.

Tra i principali strumenti anche di questa riforma, come di quella civile, che abbiamo discusso ieri, viene individuato l'ufficio per il processo, al quale vengono destinati ben 2 miliardi e 342 milioni di euro, cioè la quasi totalità dei fondi stanziati per la giustizia dal PNRR. Devo ribadire ancora una volta tutte le perplessità, mie e di Fratelli d'Italia, nei confronti di questa scelta. La giustizia, quella penale come quella civile, ha bisogno di ben altro. Ha bisogno di riforme strutturali, ha bisogno di colmare i vuoti paurosi negli organici dei magistrati (ne mancano oltre 600) e i vuoti del personale amministrativo, che, come sappiamo, ancora più ampi. Ha bisogno di ingenti investimenti per la digitalizzazione (per fortuna questi sono previsti), ma anche per la migliore organizzazione degli uffici e, in molte parti d'Italia, per la modernizzazione dei palazzi di giustizia (troppi ancora in condizioni precarie). Per non parlare dell'edilizia carceraria, perché il sovraffollamento carcerario si risolve costruendo nuove carceri e nuovi padiglioni, non abrogando di fatto la pena detentiva e liberando i delinquenti (come fate purtroppo con questo disegno di legge), né con la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha consegnato il controllo delle carceri alla criminalità organizzata. L'ufficio del processo non servirà ad abbreviare i tempi dei processi; lo sa chiunque abbia un po' di pratica giudiziaria. Tanto meno servirà a smaltire l'arretrato; per questo era molto meglio ricorrere al reclutamento straordinario di avvocati con lunga esperienza professionale e di magistrati in quiescenza, cui affidare la decisione dei procedimenti con maggiore anzianità di ruolo e minore complessità. Soprattutto, si poteva e si doveva valorizzare la professionalità di migliaia di giudici onorari, stabilizzandoli, riconoscendo loro i diritti che uno Stato di diritto riconosce a ogni lavoratore e impegnandoli nella definizione dei procedimenti di competenza del tribunale monocratico. Invece li avete mortificati ancora e continuate a mortificarli, dimenticando che, senza il loro lavoro, semplicemente la giustizia italiana avrebbe già dichiarato fallimento. Ciò premesso e ribadito che è una mera illusione credere di risolvere problemi strutturali con semplici riforme di procedura, fossero anche le più intelligenti (e queste per gran parte non lo sono), non nego che alcune soluzioni contenute in questo disegno di legge siano positive, a cominciare ad esempio dal processo penale telematico, anche se sarebbe stato necessario prevedere una maggiore gradualità nella transizione all'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali per il deposito di atti e di documenti. Così come non nego che sia positiva la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato, in modo che solo la prima notifica e la citazione a giudizio in primo e secondo grado debbano avvenire all'indagato o all'imputato, mentre tutte le altre possano avvenire al difensore. È inoltre positivo l'ampliamento del regime di procedibilità a querela e l'intenzione di restituire effettività alla pena pecuniaria, che oggi esiste solo sulla carta, visto che oscilla negli anni tra l'1 e il 2 per cento, con una perdita annuale per l'erario di circa un miliardo di euro (cioè, cari colleghi, quasi il 50 per cento dell'intero fondo stanziato dal PNRR per la giustizia, in un solo anno). Ma, a parte queste e poche altre misure positive, ce ne sono molte altre (troppe) che Fratelli d'Italia non può condividere e giudica molto pericolose. La più grave di tutte è la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità in appello e in Cassazione, attraverso il nuovo articolo 344-*bis*, con una commistione illogica e irragionevole tra un istituto di diritto sostanziale come la prescrizione e uno di diritto processuale come l'improcedibilità. Un'evidente compromesso tra le forze politiche che compongono questa spuria maggioranza, che però ha prodotto un mostro giuridico. Dovevate avere il coraggio di abrogare la riforma Bonafede. Questa era la soluzione. Quella riforma ha bloccato la prescrizione dalla sentenza di primo grado non solo in caso di condanna, ma addirittura di assoluzione. Dovevate avere il coraggio di tornare al sistema previgente, magari aumentando i termini per determinati reati di maggiore allarme o di complesso accertamento. Di questo si poteva e si doveva discutere. La soluzione di confermare la riforma Bonafede e poi limitarne l'efficacia con il correttivo dell'improcedibilità non ha alcun senso, invece. Certamente non contribuirà ad abbreviare i tempi del processo di primo grado. Infatti, basti pensare che il giudice saprà di avere a propria disposizione l'intero termine di prescrizione del reato che, come sappiamo, non è affatto breve: sette anni e mezzo per un semplice furto o per una truffa, dodici anni e mezzo per corruzione, tredici anni e un mese per peculato. Il giudice di primo grado li utilizzerà tutti, tanto sa benissimo che in ogni caso con la sentenza di primo grado la prescrizione si bloccherà e in appello si applicherà il diverso istituto dell'improcedibilità, che non terrà conto di quanto tempo è stato impiegato per decidere in primo grado. Il risultato prevedibile è una dilatazione irragionevole dei tempi dei tempi e non una loro abbreviazione, con tanti saluti all'articolo 111 della Costituzione e alla ragionevole durata del processo. Altrettanto gravi sono le conseguenze a carico delle persone offese. Sottosegretario, forse non avete ragionato su questo: le persone offese che si sono costituite parte civile per ottenere il risarcimento del danno, quando l'improcedibilità verrà dichiarata in appello o in Cassazione, vedranno anche la paralisi della loro azione in sede civile.

che impone al giudice penale sia di appello che di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato di accertare comunque il fatto ai fini degli effetti civili. Con la modifica che apportate a questa norma la decisione sarà demandata, invece, al giudice civile, con ulteriore allungamento dei tempi della decisione e con problemi di non facile soluzione - non ho trovato soluzione nel vostro disegno di legge atteso il diverso regime probatorio vigente in sede penale rispetto a quello vigente in sede civile. Faccio solo due esempi: la deposizione del danneggiato non fa prova nel processo civile, mentre fa prova nel processo penale;

Faccio l'esempio di un processo per truffa. Il giudice riterrà valide le prove assunte in sede penale in violazione dei limiti imposti invece in sede civile oppure no? Non avete regolato questo aspetto e mi preoccupa particolarmente. Altra norma molto pericolosa è quella contenuta nella lettera *i*), comma 9 dell'articolo 1, in base alla quale le procure della Repubblica potranno e dovranno individuare criteri per selezionare quali notizie di reato trattare con precedenza; con la discrezionalità di oggi! Questa sarà la vera discrezionalità, anche se nell'ambito di criteri generali dettati con legge del Parlamento. Spero Spero di sbagliarmi, ma il rischio di discrezionalità nella scelta di quali reati perseguire e quali abbandonare all'oblio e alla prescrizione è evidente. Una tale discrezionalità si pone in palese contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 12 della Costituzione. Attenzione, l'articolo 12 della Costituzione è una diretta esplicazione dell'articolo 3, in base al quale la legge è uguale per tutti; tutti siamo uguali davanti alla legge. Ebbene, questa norma viola questo elementare e fondamentale principio della nostra Costituzione. Concedere un tale potere discrezionale alle procure rappresenta pertanto una palese rappresenta pertanto una palese incostituzionalità e rischia di creare differenze inammissibili da territorio a territorio. Non è inverosimile immaginare addirittura una sorta di turismo criminale, con i delinquenti che si spostano da territorio a territorio in base alla loro specializzazione - si fa per dire - criminale, scegliendo quel territorio in cui possono contare sulla sostanziale immunità. A nulla vale obiettare che già adesso l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura procedura penale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza si tenga conto di determinati criteri di priorità. Un conto infatti è stabilire quale dibattimento abbia la precedenza rispetto ad altri che dovranno comunque tenersi; tutt'altro conto è sancire per legge quali reati le procure debbano direttamente ignorare, evitando di indagare su di essi. Vado avanti. Vado avanti. Viola certamente il diritto di difesa la previsione che, in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più componenti del collegio, il nuovo giudice possa disporre la riassunzione della pena dichiarativa solo solo se lo ritenga necessario tutte le volte in cui la stessa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione. Bastava prevedere, come abbiamo proposto (ovviamente inascoltati), che il trasferimento o il pensionamento del giudice avvenga solo al termine della trattazione dei processi assegnati. Con questa semplice misura si sarebbe risolto il 90 per cento di questo problema. Ancora, viola certamente il diritto di difesa l'inammissibilità dell'appello, che voi prevedete, quando è proposto dal difensore dell'imputato assente che non sia munito di specifico mandato successivo alla data della sentenza. Si tratta di una norma particolarmente odiosa se si considera che inciderà soprattutto sugli imputati muniti di un difensore d'ufficio, cioè sui soggetti più deboli e con maggiori difficoltà a mantenersi in contatto con il proprio difensore. Estendere difensore. Estendere l'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale minima fino a due anni - sono reati molto gravi, signor Sottosegretario, e lei lo sa ci sembra un'estensione eccessiva che in astratto potrebbe rendere non punibili reati come, ad esempio, la calunnia, la falsa testimonianza, la falsità commessa dal pubblico ufficiale, il sequestro di persona, l'usura: tutti reati che hanno una pena minima edittale inferiore a due anni nel minimo. Difficile giustificare la non punibilità di reati di tale gravità. Potrei proseguire a lungo, ma per ragioni di tempo - e ringrazio per il tempo che mi è stato concesso - mi limito a un'ultima riflessione riguardante l'ulteriore impressionante ampliamento delle pene alternative alla detenzione previsto da questa riforma. Attenzione, nessuno contesta che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, come dice l'articolo 27 della Costituzione lo cito testualmente - le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Secondo noi, però, la pena deve conservare il suo valore deterrente e di difesa sociale, ciò che viene pregiudicato dal progressivo svuotamento dell'espiazione della pena. La funzione rieducativa, infatti, a nostro avviso, deve passare attraverso l'espiazione della pena, non attraverso la sua sostanziale abolizione. Se viene meno la certezza della pena, viene meno la sua funzione deterrente e si dilata sempre di più il senso di impunità di chi tende a delinquere. Questa riforma infligge un ulteriore *vulnus* alla già blanda funzione deterrente del nostro sistema penitenziario. Questa, purtroppo, è la realtà. Fratelli d'Italia vuole processi rapidi e giusti, ma, in caso di condanna, vuole anche pene immediate e certe. Voi state andando nella direzione diametralmente opposta, mortificando ancora di più le vittime dei reati e il sentimento di giustizia degli italiani onesti. Per tutte queste ragioni il nostro giudizio su questa riforma è purtroppo negativo.

Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi, voglio fare solo alcune riflessioni stando al merito e partendo da un assunto richiamato prima dal senatore Cucca. È evidente che non esiste una riforma perfetta, ma questa è una buona riforma, che affronta

ci sono le condizioni per uscire da un'alternativa sbagliata che ha incancrenito il dibattito pubblico sulla giustizia per troppo tempo, un'alternativa sbagliata che ha schiacciato il dibattito tra una scelta che dice: «Vogliamo i processi infiniti» e una che dice:

dal disegno di legge in esame, vale a dire quella di mettere in campo le condizioni perché ci possano essere procedure e organizzazione giudiziaria che consentano tempi certi. Serve una riforma che garantisca giustizia alle vittime e un processo giusto in tempi ragionevoli, una riforma che garantisca gli imputati. Questa legge delega si

Certamente il tema dell'organizzazione giudiziaria è fondamentale, se vogliamo che davvero i processi possano essere più rapidi e la giustizia possa essere garantita a tutti. Gli investimenti di cui abbiamo parlato a lungo ieri presenti nel PNRR vanno in questa direzione. Le assunzioni, che consentono di rafforzare gli uffici del processo, gli investimenti sull'organizzazione degli uffici giudiziari, anche strutturali, gli investimenti sul digitale sono tutte scelte che possono e devono aiutare a garantire una giustizia più rapida e tempi certi, sapendo che questi sono gli strumenti concreti con cui possiamo realizzare ciò che nella norma è indicato. contiene poi altre disposizioni molto importanti. Penso, ad esempio, che la scelta di garantire tempi definiti per le indagini preliminari

serve a ridurre il carico del lavoro all'interno delle aule dei tribunali e

per particolare tenuità del fatto. Qualcuno mi deve spiegare come l'estendere la non punibilità per la tenuità del fatto possa favorire i più ricchi. Le nostre carceri sono piene di persone che hanno commesso reati davvero minori e che rimangono lì per molti anni proprio perché sono in condizioni di debolezza, non potendo avere ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, ossia

seguire, che è certamente più difficile di quella semplice che vorrebbe risolvere tutto con il carcere, magari buttando via le chiavi. Non è questa la strada che abbiamo scelto, non è la nostra. La nostra strada è quella che chiede e ottiene giustizia, applica le pene in modo ragionevole, puntando a ridurre la recidività, che il carcere produce in maniera tanto significativa, e ad aumentare la sicurezza della società italiana. Questo non significa in alcun modo dare impunità a nessuno. strumentale sostenere che la legge delega riduce la lotta contro i reati più gravi. Si è discusso, non è vero che il Parlamento non ha lavorato; si è discusso e lavorato molto in Parlamento su questo

che prevedono l'improcedibilità la dice lunga su quanto sia importante per questo Paese la lotta alle mafie. Verificheremo giustamente nei prossimi anni il funzionamento e l'efficacia della riforma. e l'efficacia della riforma. Credo si sia fatto un ottimo lavoro e si sia trovata una sintesi importante, forse impensabile solo qualche mese fa, su una materia come questa. Anche sul penale come sul civile siamo in grado di predisporre una riforma avendo gli strumenti per farla. Noi oggi siamo in grado di pensare di poter garantire più giustizia dando più garanzie agli imputati e tutelando maggiormente le vittime; una giustizia che guarda alle persone e le mette al centro. Non sono le polemiche o le contrapposizioni spesso propagandistiche che risolveranno

la pandemia, responsabile di migliaia di morti e di una crisi economica senza precedenti, ha drammaticamente messo in luce che oltre alla giustizia civile anche l'attuale architettura del sistema penale è inefficiente e produce effetti dirompenti sull'economia del nostro Paese prima ancora che sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Ci sono circa due milioni e mezzo di processi penali pendenti che sono di fatto un macigno che impedisce al sistema di funzionare. Va da sé che bisogna mettere in campo uno sforzo senza precedenti per assorbire quell'arretrato e contestualmente predisporre riforme capaci di evitare nuovi accumuli. Il *recovery fund* rappresenta un'occasione unica per poter finanziare una ristrutturazione complessiva del sistema della giustizia, per renderla efficiente e moderna. Finalmente si iniziano a coniugare riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici e accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Le modifiche che ci accingiamo a votare contengono certamente molti punti da cui partire per migliorare il nostro sistema penale. Abbiamo finalmente disponibili le risorse per investimenti attesi da anni, volti ad ammodernare anche sotto il profilo tecnologico, la lenta macchina della giustizia, a partire dalla diffusione dello strumento telematico fino alla digitalizzazione delle notificazioni. In proposito però bisogna tenere bene in mente che nessuna procedura digitale è in grado di funzionare da sola. Quindi bisognerà assicurarsi che si incrementi il personale con le competenze necessarie. Va ribadito che, a differenza degli emendamenti, le sentenze non possono essere scritte a migliaia con l'uso degli algoritmi. Quindi sarebbe opportuno implementare il numero dei magistrati e del personale amministrativo Nella sua opera «La scienza della legislazione» Gaetano Filangieri diceva che il compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza ed ai giudici ogni arbitrio. A mio avviso il processo penale italiano presenta dei vizi di fondo che risalgono alla pur meritoria riforma del 1989, aggravati dalle modifiche parziali che negli anni sono state frutto di successivi interventi legislativi. Infatti, nell'attuale sistema processuale continuano a convivere i principi di fondo di un modello processuale di matrice accusatoria e quelli che, invece, rappresentano semplicemente il retaggio di un sistema inquisitorio, nel quale la prova veniva formata nel chiuso della stanza di un giudice istruttore e manteneva la propria dignità anche al dibattimento. Nella riforma del 1989 non si è tolto nulla del sistema inquisitorio garantito, previsto dalla carta costituzionale, come ad esempio la motivazione, la prescrizione, l'appello nel merito, il controllo della motivazione in Cassazione e così via, e si è aggiunto il sistema accusatorio puro, tipo di Perry Mason, di ispirazione anglosassone, ma senza importare alcune caratteristiche peculiari di quel processo, come per esempio il verdetto popolare senza motivazione, la mancanza di un secondo giudizio di merito, il *grand jury,* anche se oggi sostituito da un incidente probatorio di rara attuazione. Il pubblico ministero, divenuto esclusivo titolare, deve svolgere le indagini secondo due ottiche diverse: il rito abbreviato, sulla cui scelta da parte dell'imputato non può assolutamente influire, che richiede la completezza della prova, e il dibattimento, dove invece la prova si deve formare *ex novo,* senza possibilità di utilizzazione di tutto ciò che si è fatto prima. Ritengo pertanto che alla fine il processo penale italiano si possa definire un ibrido e nel contempo non possa che essere uno dei più lenti, ma anche dei più garantiti del mondo. L'espansione della giustizia negoziata, il patteggiamento allargato come strumento per ridurre drasticamente i dibattimenti mi trova d'accordo, ma desta forti perplessità la passata scelta legislativa di ampliare l'area di applicazione del patteggiamento senza neppure chiedere una dichiarazione di colpevolezza, come nel modello statunitense, anzi sottoponendo poi la relativa sentenza, che è frutto di un accordo, ad un mezzo di impugnazione straordinario qual è la revisione, il che è un controsenso. controsenso. Ritengo che ci debba essere motivo di riflessione anche circa la mitizzazione del principio del contraddittorio. È vero che è un principio base del nostro ordinamento, però sarebbe necessario rafforzare il potere valutativo del giudice come arbitro delle regole del contraddittorio ed anche delle sue eccezioni, per contribuire al recupero di celerità ed efficienza del processo, evitando testimonianze interminabili senza però comprimere naturalmente le garanzie della difesa. ad esempio, prevedendo che il giudice possa disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria o da altri pubblici ufficiali, come le interminabili informative, e naturalmente lasciando poi la facoltà, a fine lettura, di rivolgere domande a chiarimento Sarebbe opportuno proporre, inoltre, l'introduzione di modalità di escussione a distanza anche di testimoni, periti, consulenti tecnici, come sperimentato nel periodo dell'emergenza Covid. Una proposta sicuramente innovativa sarebbe, infine, quella di prevedere, per la repressione dei reati di microcriminalità come furti, scippi, rapine, spaccio di stupefacenti, che mettono in crisi il senso di sicurezza dei cittadini, dei cittadini, l'intervento di un giudice che, in tempi rapidissimi, nel contraddittorio delle parti, acquisisca una prova, sempre e comunque utilizzabile, al fine di restringere al massimo, fin quasi ad annullarlo, quel periodo di tempo intercorrente tra l'originaria accusa dinanzi all'autorità inquirente e quella dinanzi al giudice. Un tempo durante il quale la vittima e il testimone rimangono, purtroppo, spesso esposti alle pressioni, alle minacce, alle intimidazioni o sottoposti ad innati e ineludibili condizionamenti ambientali. Vi sono molti altri aspetti che si potrebbero ancora prendere in considerazione per contribuire a rendere il sistema penale più efficace e snello, soprattutto in fase di impugnazione, rendendo inappellabile l'accordo su cui si fonda il patteggiamento o riducendo gli appelli meramente dilatori, attraverso la possibilità di una valutazione *in peius* delle Corti d'Appello. Infine, per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, sarebbe auspicabile eliminare il motivo del ricorso per difetto di motivazione, che finisce per trasformare il giudizio in Cassazione in un ulteriore giudizio di merito, con possibilità di rinvio e, quindi, di un infinito prolungamento dei processi. Certo, mi rendo conto che è difficile trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di speditezza e celerità del processo e quegli strumenti processuali predisposti a garanzia dell'imputato e finalizzati ad evitare decisioni ingiuste. In conclusione, però, dobbiamo dire che è un problema di scelte politiche da parte del legislatore, cui va riconosciuto il primato di stabilire se le frequenti situazioni di stallo che si verificano continuamente nel processo penale siano il necessario prezzo da pagare a momenti indefettibili di garanzia ovvero siano meri intralci e intoppi, frutto di tecniche dilatorie del tutto superflue, almeno in un'ottica di lealtà processuale tra le parti.

Oggi, come è noto, ci occupiamo del disegno di legge delega sul processo penale. Ci occupiamo, quindi, di una materia delicatissima, che riguarda la libertà e la sicurezza dei cittadini. Dico subito che non è esattamente il testo che avremmo voluto, ma è il frutto di un grande lavoro di miglioramento rispetto alla versione del ministro Cartabia, che per noi era inaccettabile. E siamo stati gli unici nella maggioranza a dirlo e a prendere una posizione netta. Questi significativi miglioramenti sono stati il frutto del lavoro del presidente Giuseppe Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, insieme al Ministro e al resto del Governo. Certo, se fossimo stati soli nell'esecutivo, l'avremmo scritta in un altro modo, ma la presenza del MoVimento 5 Stelle nell'attuale compagine governativa ha anche questa funzione, cioè quella di tenere conto della volontà popolare e del largo mandato elettorale che i cittadini ci hanno conferito nel 2018. nel 2018. Grazie al nostro impegno frenetico tra luglio e agosto scorsi, ad esempio, i termini per l'improcedibilità sono stati raddoppiati: fino a quattro anni per tutti i reati, compresi i reati ambientali, fino al dicembre del 2024; per i reati con l'aggravante mafiosa tali termini sono stati addirittura triplicati e, quindi, portati a sei anni; per tutti i reati, di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di stupefacenti, è stato eliminato il termine di durata massima. Qualcuno forse dirà che per fortuna questa non è la legge del MoVimento 5 Stelle. Bene, così sarà più facile per i cittadini capire quali valori e principi muovono le diverse forze politiche. La nostra linea è chiara da sempre ed è rintracciabile in ogni provvedimento in materia di giustizia presentato in questa legislatura in cui siamo al Governo al Governo e in maggioranza. È necessario e urgente accorciare i tempi dei processi ed è indispensabile garantire finalmente la certezza del diritto ai cittadini. Chi ha voluto vedere nella nostra linea solo o uno dei due aspetti, con l'accusa rozza secondo cui saremo quelli del "fine processo mai" dice il falso e lo sa. Questo disegno di legge reca la firma di Alfonso Bonafede perché siamo stati noi a voler riformare il processo penale, così come quello civile, mentre approvavamo la norma sulla prescrizione, che si ferma - come noto dopo la sentenza di primo grado, e mentre stanziavamo ingenti fondi per colmare i vuoti negli uffici giudiziari che si erano accumulati nel corso dei decenni. Certezza della pena e processi più brevi, grazie all'aggiornamento del procedimento e alla maggiore efficienza della macchina: queste sono le due gambe con cui rivedere la giustizia italiana. Poi, il secondo Governo Conte è caduto probabilmente anche perché queste misure, che erano state proposte sulla giustizia penale, così come altre in materia economica e sociale, non andavano bene a qualcuno. Ed ecco che una maggioranza quanto mai eterogenea, quella odierna, ha voluto rivedere le due riforme dei processi. Arriviamo oggi a votare definitivamente questo testo, ma il testo originario è a prima firma dell'ex ministro Bonafede, che ancora ringrazio per il suo lavoro.

Se in quel momento il testo non fu approvato dalle Camere è perché una forza all'interno dell'allora maggioranza faceva il controcanto continuo e spesso si comportava come opposizione interna. Posso affermare, senza tema di smentita, che oggi approviamo il testo Bonafede come emendato dal Governo Draghi, nella versione scaturita dal duro confronto con il Movimento 5 stelle, a cui facevo cenno poc'anzi. Se vogliamo dare una percentuale, almeno l'80 per cento del testo attuale si rifà al lavoro dell'ex ministro Bonafede. Aggiungo che anche la riforma del processo civile e quella del CSM erano state già approvate dal Governo precedente ed erano state bloccate dalla cosiddetta opposizione interna a interna a cui ho fatto riferimento prima. Lo rimarco per amore della verità. Per fare un altro esempio, ho sentito parlare del piano assunzionale. Ebbene, le assunzioni ordinare, che ammontano a circa 18.000 unità, a cui si aggiungono le assunzioni straordinarie, che ammontano a 21.000 unità, queste ultime previste dal PNRR, preparato dal Governo Conte II, sono state confermate dalla ministra Cartabia e dall'attuale Governo. Quindi, se oggi ci sono tanti applausi a queste porzioni della legge delega, onestà intellettuale vorrebbe che almeno una parte di questi consensi e di questi applausi fosse indirizzata a chi le ha concepite, cioè il Governo precedente, il ministro Bonafede e il MoVimento 5 Stelle che lo ha sempre sostenuto. Siamo convinti che la strada più giusta da seguire per velocizzare i processi e per una giustizia davvero giusta e ragionevolmente rapida sia ampliare gli organici dei magistrati, e del personale non togato. Ne siamo così convinti che in questi ultimi anni gli unici che su questo tema sono passati dalle dichiarazioni in Aula o nei salotti televisivi ai fatti concreti siamo stati noi del MoVimento 5 Stelle, che abbiamo varato - lo dicevo prima - il più grande piano assunzionale nel comparto giustizia da decenni a questa parte. Gli altri lo dicevano, noi lo abbiamo reso realtà. Il processo deve essere veloce, ma si deve concludere con l'accertamento dei fatti, non con un'impunità generalizzata per previsione normativa. Mandare al macero centinaia di migliaia di processi - e questo è il rischio che abbiamo corso - avrebbe significato la resa dello Stato di diritto e la morte della civiltà giuridica. Torno brevemente al punto più dibattuto di questa riforma è cioè la parte che riguarda l'improcedibilità e la prescrizione. Nel testo che viene votato oggi la prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado, così com'era previsto nella cosiddetta legge spazzacorrotti. Nel testo proposto originariamente dalla ministra Cartabia si confermava questo impianto, ma si aggiungeva - com'è noto - che in appello, decorso un termine massimo di due anni, e in Cassazione dopo un termine massimo di un anno, scattava l'improcedibilità, cioè il processo finiva nel nulla e le vittime non avrebbero ottenuto giustizia anche per reati gravissimi che destano enorme allarme sociale. Questa ipotesi per noi era inaccettabile; abbiamo alzato le barricate, sì, lo abbiamo fatto e siamo stati gli unici a farlo, perché stabilire una soglia così bassa di durata massima, cioè di due anni, in un Paese in cui il tempo di durata media in appello è maggiore - a volte anche significativamente - di due anni, in alcuni distretti di Corte d'appello, significava accettare il rischio di avere un numero spropositato di processi che sarebbero finiti nel nulla e per noi questo rischio molto concreto, come hanno ben spiegato tanti magistrati operatori del diritto, era assolutamente inaccettabile. Siamo fieri di averlo scongiurato con le modifiche che sono state introdotte grazie a noi e a cui ho fatto cenno poc'anzi. Abbiamo convinto tutti gli altri dell'Esecutivo, anche grazie alle audizioni che abbiamo chiesto in Commissione giustizia nel corso dell'esame della Camera e da queste è scaturito, per bocca di autorevoli esponenti italiani in materia di diritto e di giustizia, che c'era il rischio, con il testo originario, di creare un vero e proprio problema per la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i reati di mafia. Per l'Associazione nazionale dei magistrati, infatti, c'era il rischio di mandare al macero 150.000 processi. Tra l'altro, se non ci fossero stati i cambiamenti da noi pretesi, avremmo approvato una legge che sarebbe andata in senso esattamente contrario alle indicazioni e alle sollecitazioni che ci provengono dall'Europa, dall'Europa, che più volte - lo ricordo agli smemorati anche in quest'Aula - ha tessuto le lodi della norma sulla prescrizione contenuta nella legge spazzacorrotti. Il percorso per ottenere una giustizia giusta ed efficiente è ancora lungo, ma noi continueremo a dare il nostro apporto in modo assolutamente costruttivo, come abbiamo sempre fatto. Un apporto costruttivo ma fermo, perché non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ai nostri principi, che anzi continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione, costi quel che costi. che costi. A chi sogna di demolire tutto quello che il MoVimento 5 Stelle ha costruito in questi anni in tema di giustizia, di legalità, di rispetto delle regole e della dignità dei lavoratori, in materia di aiuto ai più fragili e agli indifesi, di giustizia sociale e redistribuzione del reddito, a tutti loro posso dire - cito il nostro presidente Giuseppe Conte - che se vorranno demolire tutto ciò dovranno passare sul nostro cadavere.

con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(per la verità non proprio unica) sull'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale è pervenuto il parere non ostativo della 5a Commissione permanente. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo la sanificazione dell'Aula si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto congiunte e quindi agli appelli nominali rispettivamente sull'articolo 1 e sull'articolo 2. Sospendo

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti in cui converrebbe tacere, per buon senso, per utilità o per esigenze personali, ma ci sono dei momenti in cui tacere sarebbe un atto da codardi da vigliacchi: questo è uno di quei momenti. La riforma Cartabia, che voteremo con convinzione è un ottimo primo passo. Come ci dice la storia, il primo passo ti toglie da dove sei, non ti porta ancora dove devi arrivare: ci toglie cioè dalla riforma Bonafede, che doveva abolire la prescrizione, ma che ha prodotto la prescrizione della riforma, e ci porta verso una dimensione nuova, di sfide importanti per il mondo della giustizia. Il dato di fatto, però, è che questa situazione viene a collocarsi nel momento più tragico della storia del potere giudiziario della vita repubblicana. Molti non hanno il coraggio di dirlo, anche tra di noi, onorevoli colleghi. Tra di noi siamo in tanti a rinunciare al gusto della verità, per paura,

non parlo dei giudici, a cui ci rivolgiamo con parole di deferente omaggio e stima, oggi, il giorno dopo l'anniversario della morte di un gigante della nostra società, quale era Rosario Livatino. Oggi, nel momento in cui ricordiamo i tanti colleghi politici, ma anche i tanti magistrati che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni, il punto vero è che il potere giudiziario è in crisi: chi lo nega, nega la realtà. Perché è in crisi? È in crisi per colpa della politica? No. La politica per anni ha discusso e litigato sulle questioni della giustizia. Diciamoci le cose come stanno, una volta per tutte: c'è stata una parte di quest'Assemblea e di quella della Camera, in particolar modo a sinistra, che ha immaginato di trarre vantaggio dalle vicende giudiziarie che riguardavano un'altra parte della politica, quella che stava nell'emiciclo di destra. È stato così: c'è una responsabilità politica della sinistra nell'aver cercato di strumentalizzare questo e della destra nell'aver risposto a questa crisi con leggi *ad personam*. C'è una responsabilità di tutti, nessuno si può tirare indietro, oggi, nel giudicare la fine di questi trent'anni di lunga guerra tra magistratura e politica. La magistratura però non ha mai avuto problemi ha sempre utilizzato ciò che avveniva in quest'Aula recuperando forza e tenendosi unita all'interno. Oggi non è più così. Perché, signora Presidente? Per tanti motivi. Il vero elemento drammatico però è che c'è una disgregazione all'interno della magistratura, che porta ad avverarsi la profezia dell'allora direttore di Radio radicale Massimo Bordin, che arrivava a definire il futuro il luogo nel quale i magistrati si sarebbero vicendevolmente arrestati. Chi di noi ha iniziato a fare politica ricordando il momento tragico e drammatico di Mani pulite non può non vedere come elemento sconvolgente il fatto che due dei personaggi del *pool*, gli unici due rimasti, oggi siano alle carte bollate tra di loro. Vi rendete conto che nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la politica avesse paura a parlare di ciò che sta accadendo in magistratura? Questo disastro del potere giudiziario oggi sta impedendo a tante donne e a tanti uomini magistrati di valorizzare ciò che essi sono e rappresentano, perché viviamo in una cappa di preoccupazione e di timore. Avverto il bisogno di dirlo qui, senza alcuna paura e senza alcun elemento di timore reverenziale. La magistratura nel 2021 ha iniziato un cammino preoccupantissimo. Perché è avvenuto questo? Per fattori politici? Perché è venuta meno la guida politica dei 5 Stelle sulla magistratura? Non lo so. Devo dare atto all'attuale Ministro degli affari esteri di aver detto parole chiare sull'uso barbaro e incivile, da parte dei 5 Stelle nel 2016, della questione giudiziaria; scuse timide scuse timide e tardive, ma pur sempre scuse, quelle del ministro Di Maio. Credo che questo tipo di scuse cancelli, almeno nel dibattito politico, il fatto che la guida del sistema della magistratura - o, meglio, del sistema della politica inerente alla magistratura - negli anni del ministero Bonafede sia stata profondamente giustizialista. Quando si diceva che giustizialismo e garantismo sono due diversi estremismi, agli amici che immaginano quella parte politica come un solido punto di riferimento del progressismo non posso che dire: "Auguri, se pensate questo". Io vengo da una cultura in cui la Costituzione è una cosa seria e il giustizialismo ne elemento di deformazione. *(Applausi)*. Al netto di questo, però, il punto fondamentale che voglio dire - e mi avvio a chiudere, signora Presidente - è che c'è un elemento chiave da affrontare. In questo momento, dopo ciò che è accaduto nel dibattito politico, sono partite, nelle dinamiche interne alla magistratura, tensioni forse mai sopite in passato, che sono esplose in una guerra oggettiva, che sta portando a indagini su indagini di magistrati contro altri magistrati. Se volete far finta di non vedere questo, fatelo pure, ma è un dato di fatto che vi riguarda, anche se fate finta di non accorgervene. E su questo c'è un punto da dire: il problema non è la separazione delle carriere, non è la separazione delle carriere, paradossalmente, ma il potere e lo strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la magistratura, che incidono nei procedimenti disciplinari dei singoli magistrati e che impediscono a magistrati bravi e di livello di fare carriera, se non sono iscritti ad alcune correnti.

laici. Bisogna avere il coraggio di dirla tutta. Il punto vero è che, se il CSM va al disciplinare giudicando sulla base dell'appartenenza alla singola corrente e non sulla base dei fatti, siamo in presenza di un problema che riguarda tutti, Chi di noi ha questioni giudiziarie a parte se le vede nelle sedi deputate. Sono intervenuto a voce e a testa alte qui

questi luoghi per affrontare le mie vicende, perché le affronto nelle sedi opportune, convinto, come sono, della limpidezza e della tranquillità del mio operato. Il punto è che riguarda anche voi. Dobbiamo riguarda anche voi. Dobbiamo prendere atto che oggi c'è un problema gigantesco di magistrati: ce ne sono alcuni straordinariamente bravi e all'altezza delle sfide del nostro tempo, che sono rinchiusi

su elementi di oggettivo malfunzionamento della magistratura, perché, quando le correnti dicono di voler stringere un cordone sanitario intorno al senatore X o Y, non si deve preoccupare quel senatore, ma il Senato. di fronte a quanto sta succedendo in questo momento, le mie conclusioni riguardano tre punti. Per esigenze di tempo, saranno tre *tweet*: i magistrati devono sentirsi liberi di fare bene il proprio lavoro, anche se non sono iscritti a una corrente; i politici devono avere il coraggio di guardare in faccia senza preoccupazioni di sorta, perché un avviso di garanzia non può bloccare una carriera; non si può continuare a parlare di nuove guarentigie. C'è un dato di fatto: le guarentigie dei parlamentari sono costituzionalmente garantite e quotidianamente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini. Se, di fronte a questo, non utilizziamo i tempi che vanno da qui al rinnovo del CSM nel luglio del 2022 per scrivere una pagina nuova, non importa chi sarà il prossimo a essere coinvolto: le vere vittime della nostra inerzia saranno la credibilità delle istituzioni e la dignità della magistratura. Non conveniva che parlassi, ma ci sono dei momenti in cui avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome è un dovere politico, civile e morale.

in mattinata ho espresso in un lungo intervento le ragioni di merito per le quali Fratelli d'Italia non può votare nemmeno questo disegno di legge Ho parlato di come non possiamo condividere questo ibrido tra prescrizione e improcedibilità, che rischia di provocare l'estinzione di migliaia di processi e risolversi in un'amnistia di fatto. Abbiamo detto che ci aspettavamo più coraggio: ci saremmo aspettati che questo Governo dei migliori avesse il coraggio di cancellare la riforma Bonafede e di tornare al regime precedente, tanto più che il 70 per cento dei reati, come sappiamo, si prescrive entro la sentenza di primo grado e la maggioranza delle prescrizioni si concentra in pochi distretti giudiziari. Sarebbe stato più opportuno intervenire in modo mirato, per risolvere le criticità che esistono in quegli uffici giudiziari e non generalizzare una soluzione che allungherà i processi, anziché accorciarli, come ho spiegato nel mio intervento in discussione generale. Avreste dovuto avere questo coraggio e invece non avete trovato di meglio che metterci una pezza peggiore del buco. Sempre in discussione generale, abbiamo criticato - e lo ribadiamo anche in dichiarazione di voto - l'introduzione di criteri di precedenza per la perseguibilità dei reati affidati alle procure, pur nell'ambito di criteri generali stabiliti con legge del Parlamento. È una palese violazione degli articoli 112, che prescrive l'obbligatorietà dell'azione penale, e 3 della Costituzione, della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, secondo il quale tutti siamo uguali davanti alla legge. Avete introdotto una discrezionalità incostituzionale, che rischia di portare addirittura a un turismo criminale, a seconda dei criteri che verranno stabiliti procura per procura. Non Non condividiamo inoltre l'appello del difensore dell'imputato assente soltanto se munito di mandato in data posteriore alla sentenza: un burocratico formalismo inventato solo per impedire l'esercizio del diritto di difesa, che penalizzerà inevitabilmente i più deboli e i meno garantiti. Neppure condividiamo la regola del giudizio di appello non partecipato, salvo diversa richiesta dell'interessato: è un pregiudizio verso il principio dell'oralità, che è un cardine della nostra civiltà giuridica, che state demolendo

Non condividiamo soprattutto la sostanziale abolizione della pena detentiva e della certezza della pena, che avete trasformato in certezza dell'impunità. Fratelli d'Italia è per le massime garanzie nel processo, ma è anche per il massimo rigore nell'esecuzione della pena. Voi state facendo esattamente il contrario.

e quella della responsabilità civile dei magistrati, che è un privilegio medioevale. Tutti rispondiamo dei danni che provochiamo, tranne i magistrati, che rispondono soltanto indirettamente e nel limite massimo di sei mensilità del loro stipendio: è una vergogna soltanto italiana, che voi ovviamente non avete il coraggio di affrontare, come non lo avete di affrontare la riforma del CSM per fermare finalmente la lottizzazione delle cariche più importanti tra le correnti della magistratura. Non avete nemmeno il coraggio di parlare della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, senza la quale non si avrà mai un giusto processo. Tutto questo lo realizzate

Cara Ministra Cartabia, il suo Governo dei migliori ha trasformato il Parlamento in una scatola vuota, nel silenzio

ma addirittura la dialettica democratica e il confronto parlamentare. Vi ricordo, cari signori del Governo, che l'Italia è una Repubblica parlamentare e che la sovranità appartiene al popolo, che è rappresentato dal Parlamento. Vi siete scordati questo piccolo particolare: andate avanti solo a colpi di fiducia, vi mettete d'accordo fra di voi al chiuso delle vostre stanze e ve ne fregate dei principi della Costituzione, sui quali avete votato. Per queste ragioni, non siamo mai stati più convinti di ora nell'esprimere non soltanto il nostro voto contrario a questa ennesima fiducia, ma tutta la riprovazione di cui siamo capaci per questo modo vergognoso di gestire la Cosa pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, la discussione su questa importantissima riforma - e non poteva che essere così - ha riportato il dibattito su un tema molto, molto importante, spesso agitato e spesso agito in maniera impropria: il tema del garantismo, dello stato di diritto, di ciò che ci distingue

schieri tra garantismo e giustizialismo: lo schierarsi è tra impunità e giustizialismo, perché dovremmo essere tutti garantisti; è una precondizione del riconoscersi in questa Costituzione. Naturalmente, poi, dobbiamo vedere quando si fanno garantismo di maniera o giustizialismo a correnti alternate, perché sono ben pochi coloro che, tra gli esponenti politici,

che, insieme alla ragionevolezza, oltre ad essere ovviamente principio costituzionale, non è una via di mezzo tra appassionanti tesi e battaglie: l'equilibrio e la ragionevolezza sono una cifra, che

stiamo decidendo della libertà e, delle sorti dei nostri cittadini, che in quel momento incontrano lo Stato con la sua potenza, indipendentemente dal censo (e non vorremmo ovviamente che questo fosse una scriminante). Lo incontrano le persone offese, chi ha subito un danno o un offesa, e infine i cittadini, perché la sentenza è pubblica ed è nel nome del popolo italiano esattamente per questo motivo. Noi siamo per le regole nel processo e siamo perché questo equilibrio venga garantito e assicurato. Non abbiamo alcuna nostalgia per quei tempi in cui un processo, come ad esempio quello sulla strage di Piazza Fontana, poteva essere spostato da una parte o dall'altra, utilizzando la *legitima suspicione*: non abbiamo nostalgia di quel tipo di magistratura, che non poteva essere indipendente.

e proposto la valutazione della professionalità, anche tenendo conto dell'eccessiva discrepanza tra richiesta di rinvio a giudizio e assoluzioni. Ciò è nella riforma del processo penale, perché è previsto che si possa avere un rinvio a giudizio solo in presenza di una ragionevole previsione di condanna. Proponiamo inoltre un'Alta corte per i giudizi disciplinari dei magistrati in grado d'appello.

all'equilibrio, siamo quelli che hanno introdotto gli ecoreati, che danneggiano la salute dei cittadini, e hanno ripristinato il falso in bilancio, che è collegato alla corruzione.

Con tempi eccessivamente lunghi, si lascia spazio a una gogna mediatica e il principio di non colpevolezza viene sostituito da una presunzione di colpevolezza. Quando c'è il cortocircuito mediatico, c'è un tema che ha a che vedere con le indagini e la sovraesposizione delle procure.

per esempio, della questione che riguarda l'iscrizione al registro delle notizie di reato, che è un punto nevralgico delle garanzie per chi viene sottoposto a un processo che può addirittura essere retrodatato. Si tratta di un intervento importantissimo. Non si è parlato del fatto che, oltre all'ampliamento dei riti alternativi, si può patteggiare una pena sostitutiva fin dalla fase del processo, senza aspettare anni, quando diventerà esecutiva.

Dobbiamo chiudere definitivamente una stagione che ha portato solo mali alla giustizia. C'è il regolamento di conti tra i poteri dello Stato. il tema dell'equilibrio - e torno a questa parola - tra i poteri dello Stato. Tuttavia, non è inaugurando una nuova stagione di regolamento di conti che lo affrontiamo lo affrontiamo con interventi incisivi, che infatti non sono indolori, perché - come vedete - provocano dibattiti e contrapposizioni che dobbiamo ascoltare.

Siamo quelli che hanno lavorato per trovare una soluzione, la più condivisa possibile. Anche questo è senso di responsabilità, nell'ambito di tutte le soluzioni tecniche che erano state prospettate. In In definitiva, il luogo delle riforme è il Parlamento, quindi non è un regolamento di conti in altre piazze; sì alle riforme e agli interventi giusti e necessari, qui ed ora. da qui infatti, dal Parlamento, che parliamo ai cittadini, alla loro vita, alle loro garanzie, ai tempi della loro vita e alla loro dimensione umana esistenziale e di cittadini in Europa e in Italia. Da qui, da questo Parlamento, stiamo nell'Europa e guardiamo ad essa a testa alta, non solo per fare i compiti che ci vengono prescritti prescritti collettivamente, ma perché noi siamo l'Italia e sul diritto, sulle garanzie e sulla Costituzione sappiamo come si fa e abbiamo qualcosa da dire. Grazie,

Vorrei rasserenare il senatore Renzi (che però non vedo più in Aula), perché ho presentato

cui si preveda il sorteggio, si possano trovare soluzioni che diminuiscano nel CSM il potere delle correnti nella magistratura. Invito quindi il senatore Renzi a firmare eventualmente il disegno di legge, che è già calendarizzato, e il Gruppo Italia Viva ad appoggiarne l'*iter* per portarlo all'approvazione. Detto questo, sono d'accordo con il senatore Renzi: quanto ci apprestiamo ad approvare oggi costituisce sicuramente una base di partenza e non di arrivo per accelerare i processi e diminuirne il numero, senza depotenziare le garanzie difensive e tutelando quindi le vittime. Certo, si riducono alcuni momenti di stallo del processo, dobbiamo dare atto di questo; si estendono le tipologie dei reati per i quali è prevista la citazione diretta davanti al tribunale monocratico; si amplia il numero dei reati procedibili a querela; si promuove una digitalizzazione del processo penale per renderlo più moderno, introducendo l'obbligo di utilizzo delle modalità digitali; si ampliano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e questo avrà certamente una ricaduta positiva anche sul sistema carcerario, evitando sovraffollamenti. A tal proposito, scusate l'inciso, ma, signora Ministra, mi pare che sia inconcepibile quanto avvenuto nel carcere di Frosinone, dove un detenuto è entrato in possesso di un'arma, ha sparato ad altri detenuti, ha minacciato agenti di polizia penitenziaria (che - lo ricordo - non possono avere armi con loro all'interno degli istituti) e poi ha chiamato - attraverso un cellulare, anch'esso posseduto illegalmente - il proprio legale. Torniamo però al tema che ci occupa. Discorso a parte merita la nuova disciplina sulla prescrizione, da molti percepita come un cardine della riforma. Non sono completamente d'accordo al riguardo. Malgrado non condivida la nuova disciplina dell'improcedibilità che si pone come rimedio definitivo per l'eccessiva durata dei processi, comprendo però le ragioni di mediazione politica sul tema e ritengo tutto sommato accettabile la soluzione prospettata, che prevede proroghe ulteriori in caso di complessità con tempistiche ulteriori in caso di delitti commessi per finalità di terrorismo, eversione, banda armata, associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza sessuale aggravata e altri reati, come quelli contro la pubblica amministrazione. Si auspica che, come previsto da un ordine del giorno approvato in Commissione, tra questi reati possa rientrare, con un successivo intervento legislativo, anche il disastro ambientale. Si ricorda che resta esclusa, ma per la disciplina già vigente, l'applicabilità dell'improcedibilità per i delitti puniti con l'ergastolo e questo è tranquillizzante. Nei vari tavoli a cui ho partecipato, ho molto insistito sull'opportunità di queste proroghe e sulla necessità di mettere al riparo i processi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, specialmente per reati di mafia e terrorismo, perché sono processi assolutamente diversi, in cui non bisogna provare soltanto la responsabilità, ma spesso ricostruire un contesto ambientale, e quindi sono già per definizione complessi. Ho accolto con favore, quindi, la disposizione transitoria che prevede che le nuove norme si applichino solo nei procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 1° gennaio 2020. C'è stato un lavoro lungo, molto complesso, in seno alla maggioranza, in riunioni e confronti nei quali si sono toccate con mano le profonde divergenze (di cui ha preso atto) che animano i rapporti tra forze politiche così eterogenee per visione e valori. canto mio, ho cercato in ciascuna occasione - sì, lo ammetto - di alzare un po' l'asticella dell'accordo. Nei tanti anni in cui ho svolto la professione di magistrato, mi sono infatti convinto che al sistema giustizia occorra un cambiamento drastico, che ridefinisca radicalmente il sistema processuale: fare una scelta decisa tra quello accusatorio e quello inquisitorio garantito che c'era prima. Ho preferito non presentare emendamenti, così come hanno fatto altri colleghi, perché, apprezzate tutte le circostanze, credo che sia importante non rallentare il percorso della riforma, che è assolutamente necessaria al Paese. Con spirito istituzionale, quindi, voterò insieme al mio Gruppo la fiducia al Governo, senza rinunciare però alla sincerità. C'è ancora molto da lavorare per poter parlare di una svolta innovativa e di una vera e propria riforma. Ci sono alcuni aspetti problematici, come ad esempio l'aver esteso la tenuità del fatto a reati come la falsa testimonianza, l'omicidio colposo o il sequestro di persona. Aggiungo che aver previsto che sia il Parlamento a dettare i criteri generali di priorità per l'esercizio dell'azione penale alle procure costituisce un *vulnus* (come sa bene) al principio costituzionale della separazione dei poteri, che non è solo costituzionale, ma risale a Montesquieu. A questo punto, quindi, ci attende un fondamentale lavoro, dopo l'approvazione della delega, in un rapporto dialettico sano tra Governo e Parlamento, che mi auguro riguardi tutte le altre questioni che stiamo affrontando. A tal proposito, mi sia consentita un'ulteriore riflessione. La pandemia ha stravolto nel profondo il nostro Paese: nel corso di pochi mesi, è cambiato il nostro modo di pensare alle priorità, di interpretare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e di vivere il nostro quotidiano. Molte sono le domande cui le istituzioni devono dare risposta, mentre curano migliaia di persone, tentano di risollevare la nostra economia e intraprendono un difficile percorso per affrontare le sfide globali per molte di queste domande non esiste già una risposta, ma bisognerà trovarla e bisognerà farlo insieme. Non è irrilevante il metodo, che lei stessa ha annunciato, attraverso il quale devono maturare queste risposte:

Credo sia opportuna un'ulteriore riflessione. Nel momento in cui la democrazia parlamentare che abbiamo sin qui conosciuto subisce cambiamenti sostanziali e decisivi a Costituzione invariata, pur comprendendo le ragioni di contesto, ritengo preoccupante la riduzione sostanziale del ruolo del Parlamento nel processo decisionale. Capisco la tentazione di accelerare la procedura parlamentare anche attraverso lo strumento tecnico della fiducia, anzi di due fiducie su ogni articolo, come ho appreso. Capisco e condivido l'esigenza della tempestività imposta dalla crisi. Capisco e condivido la paura di mancare l'opportunità innescata dal *recovery plan*. Allo stesso tempo, però, trovo molto difficile, se non addirittura pericoloso, accettare che il Parlamento, anche se in un solo ramo, si limiti a ratificare decisioni, piuttosto che ispirarle. Ciò premesso, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali.

il presidente Renzi oggi ha posto una questione che non possiamo far finta di dimenticare. Senatrice Rossomando, lei ha fatto riferimento alla questione tra garantismo e giustizialismo. non sono garantista come modo di dire: credo che il garantismo sia applicazione delle regole, qualunque sia il risultato,

però il Ministro della giustizia, ritenendo di poter rispondere a tutte le questioni con una bozza di legge per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura: non aveva capito nulla.

Quella magistratura, però, era realmente indipendente, aveva fatto certamente salti di qualità, rispetto a una professionalità che era stata conquistata sul campo, e aveva avuto appunto la possibilità di resistere al terrorismo, in quegli anni, significava resistere con processi senza leggi speciali, e quelle conseguenze le abbiamo ancora oggi. oggi. Certamente lo sforzo che ha fatto il Governo è enorme, ma bisogna cominciare a valutare le questioni. Certamente è stato introdotto un maggiore equilibrio tra le parti processuali, avvocati e pubblico ministero, nella fase delle indagini. Signor Ministro, faccio parte di Forza Italia. Credo nella separazione delle carriere, ma nemmeno questa ci garantirà un'effettiva parità, perché il pubblico ministero avrà comunque strumenti e possibilità di utilizzarli ben diversi dall'avvocato.

È normale? È conseguenza del nostro codice? Non credo. Allora, c'è qualcosa che non funziona. non funziona. Quelle che metterò in evidenza sono alcune questioni che ho già sollevato per ben otto anni: il controllo giurisdizionale al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. L'ho presentato all'epoca del Governo di cui faceva parte il ministro della giustizia Orlando e non l'abbiamo fatto.

nel 2013, quando abbiamo detto che si poteva applicare alla Commissione per la verifica dei poteri un regolamento diverso, perché quello era un organo paragiurisdizionale e non giurisdizionale, come invece ha detto la Corte costituzionale

dell'azione penale, che solo il Parlamento può indicare, nemmeno il Consiglio superiore della magistratura? Chi ha detto che questi criteri generali dovevano essere sviluppati all'interno delle singole procure?

Io non sono di quelli che vivono della voglia di galera per gli altri. È questa la ragione, caro Ministro, di tutta questa situazione che non funziona. Infatti nel momento in cui abbiamo introdotto pene altissime, per cui il processo non si prescrive, perché questa follia di Bonafede di prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Lei sa quando arriva la sentenza di primo grado?

che tutti quelli che avranno processi più lunghi, avranno poi la possibilità di rivolgersi allo Stato per essere risarciti della violazione sotto il profilo dell'irragionevolezza dei

né più, né meno modulato secondo i tempi fissati dalla Corte europea sotto il profilo della durata dei processi. Quando chiesi ad Anna Finocchiaro

e qui è il problema e capisco benissimo - le ragioni politiche che hanno portato a questo. Ha ragione il nostro amico Alberto Balboni: nel momento in cui si mette in evidenza la contraddizione,

perché la nostra vita è retta dalla civiltà giuridica della legge che regola i rapporti tra i cittadini. Signor Presidente, l'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha determinato l'insorgere di gravi rischi, ma anche di inedite potenzialità di ricostruzione del sistema della giustizia penale, che resta esposta ad un forte stress a causa della rigidità dell'apparato organizzativo intero e delle procedure. Il fenomeno epidemico si colloca all'interno di uno scenario storico ordinamentale della giurisdizione penale già attraversato da una profonda crisi di effettività ed autorevolezza, le cui ragioni sono ben note: la smisurata quantità di notizie di reato, sproporzionata rispetto alla capacità di trattazione; l'ipertrofia dell'inchiesta, che in assenza di pregnanti controlli del giudice è divenuto il baricentro mediatico del rito e dalla quale sorge il prevalere delle ansie securitarie e il pregiudizio di colpevolezza dell'indagato; la ridotta utilizzabilità dei riti semplificati di tipo premiale, che avrebbe dovuto dare respiro al processo accusatorio; l'irrazionale proliferazione dei rimedi impugnatori in difetto di filtri efficaci; le cadenze temporali asfittiche e non regolamentate della procedura. La risposta idonea a restaurare la cultura della giurisdizione e le linee fisiologiche del giusto processo, i cui valori sono incisivamente scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione, consiste nell'implementare, come nel testo in esame, l'efficacia della giurisdizione penale attraverso un'opera di ricostruzione dei momenti topici della verifica dell'ipotesi di accusa e dell'accertamento della verità, nel rispetto delle garanzie, lungo itinerari più semplici, trasparenti, celeri ed efficienti. Occorreva quindi, come in questo caso, con grande sforzo, coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie. L'inchiesta investigativa, in assenza di pregnanti controlli del giudice per le indagini preliminari, è diventata l'effettivo baricentro del rito. Da essa spesso sorge, anche per il ricorrente intreccio di relazioni tra uffici di procure ed organi di stampa, il prevalere nella collettività del pregiudizio di colpevolezza dell'indagato, inesorabilmente colpito dalla gogna mediatica, con il conseguente rischio che prevalgano logiche di chiusura corporativa opposte alla linea costituzionale dell'attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione. Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una giusta serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, misure che sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata. In particolare, fondamentali sono i principi e i criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, incidendo sui termini di durata delle indagini, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla, sia agli effetti dell'iscrizione, prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano sia civile che amministrativo; sulla fase conclusiva delle indagini, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare limitandone la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore, nel massimo, a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento, prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione. Incide in particolare per quanto riguarda la regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una ragionevole previsione di condanna; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili. principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Nel giudizio abbreviato il Governo interverrà sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Dovrà prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. L'articolo 1, al comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il Governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito. Dovrà prevedere inoltre che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Sulla scorta di questi dati, che rappresentano un punto di sintesi fondamentale per il prosieguo in un settore quale quello della giustizia penale, che ha riflessi sociali importantissimi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, atteso che si è davvero voluto intervenire con misure non più rinviabili, volte al recupero di efficienza del sistema procedurale.

onorevoli colleghi senatori, devo dire che ho avuto un iniziale smarrimento ascoltando il primo intervento, quello del *leader* di Italia Viva Matteo Renzi. Non voglio assolutamente sindacare sul coraggio che si autoattribuisce dichiarandosi l'unico uomo della galassia ad avere il coraggio, appunto, di parlare di magistrati e magistratura, ma temo che abbia confuso l'ordine del giorno, perché oggi parliamo della riforma del processo penale, non della riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi)*. Detto questo, Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare reca la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Reputo questa una riforma importantissima, che persegue alcune finalità come, ad esempio, la deflazione del processo penale e la sua accelerazione, la digitalizzazione; maggiori garanzie difensive e maggiori tutele per la vittima e l'implementazione della giustizia riparativa e poi la prescrizione e l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

del Governo Conte, Bonafede, e ad essa si collegano la riforma della giustizia civile e quella dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura.

il taglio della prescrizione, così come intesa dal Movimento 5 Stelle, è stato inserito in un disegno molto più grande e più complesso, per accelerare i tempi della giustizia, composto da migliaia di assunzioni nel comparto della giustizia, a partire dall'ampliamento dell'organico della magistratura, passando per quello dei tribunali e terminando con quello delle carceri. A ciò aggiungiamo anche il finanziamento di ingenti somme, destinate alla geografia giudiziaria e a quella carceraria. Voglio chiarire un punto: non stiamo votando una riforma scritta in fretta e furia dal Governo Draghi, perché la riforma Bonafede era da cestinare.

l'Italia aveva già tre riforme della giustizia pronte, perché erano già state approvate dal Consiglio dei ministri: quella della giustizia civile, che abbiamo già approvato, quella della giustizia penale e quella del CSM.

epocale per quel che riguarda le assunzioni di personale nel comparto della giustizia. Essa è epocale, perché non ci sono precedenti di un piano ordinario di assunzioni di circa 18.000 unità, al quale si aggiunge il piano straordinario,

che l'impianto della prescrizione, inteso dal MoVimento 5 Stelle e dal ministro Bonafede, è rimasto quello ideato nel 2020, per quanto riguarda il primo grado.

Con più personale, infatti, aumenta l'efficienza della giustizia ed ecco che il tema della prescrizione si sgonfia, perché i processi vedranno una fine e la macchina della giustizia funzionerà meglio. Siamo stati e rimaniamo gli unici a voler affermare un principio sacrosanto: l'inefficienza non può tradursi mai in impunità. Tornando quindi alla parte più dibattuta, dal punto di vista politico, ovvero la disciplina dell'improcedibilità, così come è stata proposta dal Governo, al MoVimento 5 Stelle non poteva andare bene, perché prevedere il limite di due anni in appello per dare luogo all'improcedibilità, facendo finire oggettivamente nel nulla il processo penale, in un Paese in cui la durata media supera il termine dei due anni, per noi vuol dire incentivare e sollecitare il ricorso in secondo grado, ingolfando così le Corti d'appello e ottenendo l'effetto contrario a quello che deve essere lo scopo della riforma e cioè accelerare i tempi della giustizia. Cosa abbiamo fatto, noi? Abbiamo chiesto subito un implemento di audizioni, dalle quali sono emersi due campanelli d'allarme. Il primo è il rischio di un problema di sicurezza nazionale per i reati di mafia; il secondo, conseguente, è il rischio di mandare al macero 150 processi penali. Ci siamo fatti carico di queste preoccupazioni, nella quasi totalità del silenzio della politica. Dico quasi, perché una voce si è sentita - purtroppo, aggiungo - quella del segretario della Lega Matteo Salvini, il quale ha affermato che la riforma non andava toccata, ignorando completamente l'allarme che veniva lanciato da chi della lotta alla mafia ha fatto una ragione di vita, cioè i magistrati antimafia, Presidente. Questo ci ha meravigliato, perché da chi è stato Ministro dell'interno, ovvero Ministro della sicurezza nazionale, ci si aspetta un altro atteggiamento, sicuramente più sensibile ai temi della lotta alla criminalità organizzata. Le mafie non si combattono con le felpe e con gli slogan. poi denunciare il comportamento di Forza Italia, che invece approfittava della confusione tentando maldestramente l'inserimento di un emendamento sull'abuso d'ufficio, tentativo sventato sempre dal MoVimento 5 Stelle.

Cos'è che abbiamo fatto, sempre noi? Abbiamo chiesto e ottenuto che per tutti i reati, compresi i reati ambientali *(Commenti)* - ascoltate, colleghi fino al dicembre 2024 i termini per l'improcedibilità in appello, in determinate condizioni, venissero raddoppiati a quattro anni (non più due). Per i reati di mafia, sempre noi abbiamo ottenuto il prolungamento del termine di improcedibilità che non è più di due, ma di sei anni. E ancora sempre noi, perché noi siamo il MoVimento 5 Stelle *(Applausi)*, perché per noi lo Stato non può dire a chi attende giustizia che è suonato il gong e che per questa volta non se ne fa nulla, abbiamo ottenuto che per tutti i reati di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, di terrorismo,

Prego, senatore Lomuti, continui, se gentilmente l'Assemblea permette a un collega di terminare il proprio intervento. LOMUTI *(M5S)*. Grazie, Presidente, ma non li sento, Concludo. Siamo grati alla ministra Cartabia per averci dato l'opportunità di riaprire un dialogo costruttivo, prima di andare in Aula con questa riforma. Ma dobbiamo precisare che su questi aspetti questa non è la nostra Non abbiamo mai pensato che il testo non potesse essere migliorato e così abbiamo fatto. Il MoVimento 5 Stelle ha alzato le barricate perché non possiamo transigere sui processi per mafia e terrorismo; oggi, grazie al MoVimento 5 Stelle, questi processi non si dissolveranno nel nulla. *(Applausi).* Se per questi risultati veniamo etichettati come giustizialisti, rispondiamo che bisogna smetterla di dire menzogne ai cittadini. Cari colleghi, senza legalità non ci può essere sviluppo nei territori. Signora Ministra, c'è ancora molto da lavorare e lo faremo nei decreti attuativi con questo spirito. Nel ringraziare il ministro Alfonso Bonafede, il nostro Ministro, e il presidente Giuseppe Conte *(Applausi. che hanno messo in campo per migliorare aspetti importanti di questa riforma, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. Questa riforma reca fortissima la cifra del Governo Draghi. Da un lato autoritarismo e accentramento del potere, che si sono manifestati nel non consentire al Senato e neanche alla Camera di modificare alcunché e soprattutto nell'indicazione precisa di normalizzare la magistratura, perché, come sapete, viene previsto che sarà la politica e quindi sempre il Governo, che detta legge anche nel Parlamento, a indicare quali saranno le priorità per le procure e quindi sostanzialmente quali reati perseguire e quali invece lasciar correre. Dall'altro lato, la cifra ancora più marcata di questo Governo è l'elitarismo, la difesa degli interessi della casta, dei colletti bianchi, dei politici, degli amministratori, dei ricchi sostanzialmente, che si manifesta nelle sacche di impunità previste da questa riforma. L'elemento macroscopico è l'improcedibilità che consentirà a tutti coloro che se lo potranno permettere attraverso cavilli e buoni avvocati di prendere tempo e di arrivare all'improcedibilità, magari anche dopo essere stati condannati in primo grado. Basterà tirarla abbastanza per le lunghe e magicamente, dopo due anni in appello o un anno in Cassazione, ci sarà l'improcedibilità. Anche nel caso in cui ci fosse la proroga, è sempre pronto il cavillo perché il provvedimento dovrà essere motivato per la particolare complessità del giudizio, sarà ricorribile in Cassazione e, quindi, chi non ricorrerà in Cassazione? In quella sede si discuterà non della colpevolezza o dell'innocenza, ma della sufficiente motivazione per giustificare la proroga sulla base della

Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti

14a e questioni regionali. Le predette Commissioni sono autorizzate a convocarsi al fine di consentire alla 1a Commissione di riferire all'Assemblea nella seduta di

1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Allegato B).* Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge. Indìco la votazione dell'articolo 2,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 Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Lonardo).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale del disegno di legge al nostro esame avrà luogo nella seduta di domani.

Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire ieri perché ricorreva il trentunesimo anniversario del barbaro omicidio del giudice

Salvini ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo, Renzi invece vorrebbe promuovere un *referendum* abrogativo. Il ritornello ripetuto fino alla noia è che il reddito andrebbe, a loro dire, a mafiosi, delinquenti o a gente che non ne avrebbe diritto; tuttavia i dati ufficiali smentiscono categoricamente queste che, dal nostro punto di vista, sono delle menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per cento dei beneficiari è risultato irregolare. Io sarei davvero felicissimo se si registrassero tassi di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente a cittadini e imprese, ma di cui non si parla mai perché non sono stati approvati e promossi dal MoVimento 5 Stelle. I detrattori affermano che per colpa del reddito cittadinanza non si troverebbero lavoratori stagionali,

i contratti per i lavoratori stagionali a maggio del 2021 sono stati 148.000, molti più di quelli che si sono registrati nel 2020. Questo è abbastanza

particolarmente grave che si faccia questa propaganda a discapito di gente fragile, di nostri connazionali in situazione di difficoltà, che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato può e deve dare loro, quindi davvero ci aspettiamo che questa ignobile propaganda abbia termine al più presto possibile Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per richiamare l'attenzione sua e di quest'Assemblea rispetto all'ennesimo atto di aggressione nei confronti di personale medico e sanitario. avvenimenti di questi ultimi giorni occorsi nella mia provincia, Siracusa, dove a Portopalo un collega è stato violentemente aggredito da due facinorosi che lo hanno scaraventato a terra provocandogli una lussazione della spalla; inoltre, in una guardia medica, un paio di giorni fa un soggetto violento ha colpito con una testata un operatore sanitario perché gli rifiutava l'ingresso.

comunque norme per aumentare la tutela del lavoro dei sanitari. Noi medici e tutti gli operatori sanitari andiamo al lavoro per salvare le vite. Non vorremmo assolutamente rimetterci la nostra, così come vorremmo non accadesse in tutti gli altri settori del

organizzato questa manifestazione, che si è tenuta domenica scorsa in piazza Duomo nella città aretusea. È stata una manifestazione silenziosa, nel corso della quale, però, abbiamo espresso il concetto ispiratore di questa manifestazione: